Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, quello che ci accingiamo ad esaminare, il disegno di legge *made in Italy*, è certamente un provvedimento cardine, soprattutto per la politica industriale del nostro Paese, nostro Paese, strutturale e strategico per tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo, il *made in Italy*. Il disegno di legge n. 958 reca «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023, trasmesso il successivo 11 dicembre e assegnato nella stessa data alla 9a Commissione in sede referente. Il disegno di legge consta di 59 articoli. L'articolo 1 chiarisce che le norme in esame sono volte a valorizzare le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, ai fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale. Nell'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge e ai sensi di quanto prevede l'articolo 2, le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a orientare la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, della promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e della eco-innovazione, dell'inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile. L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy*, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana. L'articolo 4, modificato durante l'esame parlamentare alla Camera, istituisce, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica, e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidati un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di 15 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo del 2000, destinato al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili. L'articolo 6 prevede per l'anno 2024 la concessione alle *startup* innovative e alle microimprese dei Voucher 3I-Investire In Innovazione, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2019 per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto. L'articolo 7, inserito alla Camera dei deputati, obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquant'anni o per il quale sia possibile dimostrare

e i motivi che impongono la medesima cessazione. In caso di notifica, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al Mimit di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Per i marchi che risultano non utilizzati da almeno cinque anni, il Mimit può depositare a proprio nome domanda di registrazione del marchio. Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero. L'articolo 8, come modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno. sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), promuova lo sviluppo della certificazione della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive dell'industria della prima lavorazione del legno. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Il comma 3, come modificato dalla Camera, reca inoltre norme di coordinamento normativo in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali. L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il MASAF, al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. L'articolo L'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il Mimit promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame alla Camera, stanzia 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. L'articolo 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da sessanta a sette giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista L'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

La norma consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti in navigazione in acque territoriali straniere, di attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI). L'articolo 15 prevede L'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mimit, delle aree di interesse strategico nazionale. prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità. L'articolo 17 istituisce presso il Mimit una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida. L'articolo 18, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera, comma 1 istituisce il percorso liceale del *made in Italy,* che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. L'articolo 19 dispone la costituzione della Fondazione denominata Imprese e competenze per il *made in Italy*. La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy,* di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. L'articolo 20 istituisce l'esposizione nazionale permanente del *made in Italy,* affidandone la cura e la gestione alla Fondazione Imprese e competenze per il *made in Italy.* L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il MASAF, nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. L'articolo 22 consente agli istituti e ai luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza, di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

c'è un'espressione in inglese, quell'idioma tanto amato da uno dei parlamentari della maggioranza, che caratterizza uno dei Ministeri del Governo Meloni, ed è il *made in Italy*. È un'espressione utilizzata dagli anni Ottanta che caratterizza e racchiude il patrimonio culturale, la filosofia produttiva e l'impronta di qualità del nostro Paese.

la vocazione manifatturiera del nostro Paese è talmente apprezzata nel mondo da far considerare il *brand made in Italy* uno dei più importanti a livello globale. In concreto, il luogo in cui viene prodotta l'eccellenza, la *delivery,* influisce notevolmente e profondamente sulla sua essenza. Ogni Regione possiede una peculiare identità culturale e strutturale, che sostanzialmente si riflette sul prodotto finale. Sotto questo profilo, signor Presidente, l'Italia detiene uno dei patrimoni storico-culturali più importanti al mondo. La sua lunga storia, unitamente alla peculiarità del suo settore agroalimentare, la rendono uno dei Paesi più visitati al mondo. L'indicazione *made in Italy* può essere applicata ad un prodotto o quando questo viene

viene apposta l'etichetta del Paese di origine. È proprio su questo punto che bisogna porre la massima attenzione, perché la robustezza del *made in Italy* risiede, infatti, proprio nell'originalità, nella qualità, nella perfezione e nel pregio delle creazioni italiane in diversi settori, tra cui moda, arredamento, alimentari, meccanica, artigianato e anche nella fornitura della posa in opera. Presidente, mi chiedo e vi chiedo se, a fronte dell'incremento esponenziale dei casi di contraffazione e di plagio del nostro *brand*, effettivamente le risorse messe a disposizione non siano esigue. Ebbene sì, signor Presidente, sono esigue, tratti di un provvedimento in cui il *made in Italy* è proprio il vessillo. Lo dico senza mezzi termini: non solo le risorse sono esigue, ma vengono spostate da un capitolo all'altro con il classico gioco delle tre carte, dove però tutti perdono. Eppure, Presidente, mentre noi ci troviamo nella sacralità di quest'Aula, sappiamo - e questo lo certificano i *report* della Guardia di finanza - che ci sono migliaia di aziende nel mondo che sfruttano illecitamente il marchio del *made in Italy* e per tutta risposta il Governo Meloni propone un testo che sa unicamente di zibaldone leopardiano, dove si parla di tutto e di niente, pensato male e scritto anche peggio. Al netto di questa sterile operazione elettorale - l'ennesima, per dire la verità, Presidente - ci si trova ancora indietro, totalmente inerti innanzi alle minacce che provengono dai *competitor* internazionali e da chi cerca di scipparci il nostro orgoglio nazionale. C'è un tema, poi, che va affrontato ed è quello della competitività, perché al netto delle minacce truffaldine è anche vero che la nostra industria deve evolversi e per essere competitivi bisogna essere digitali. La digitalizzazione, quella fortemente voluta e sostenuta dal Governo di Giuseppe Conte, è essenziale per rimanere ancorati a questo villaggio globale, perché restarne fuori, anche minimamente, non comporta che svantaggi sia per la vendita sia per la pubblicità. Urgono quindi un cambiamento di passo, un incremento delle infrastrutture digitali e soprattutto un maggiore intervento dello Stato per far sì che queste aziende possano attaccare la spina ai processi produttivi capaci di incrementare l'efficienza e l'efficacia del nostro tessuto imprenditoriale. Le aziende italiane hanno la necessità di avere un'infrastruttura di rete che permetta loro di essere competitive. Parlare di fibra ottica sembra normale per chi vive in complessi cittadini o in aree industriali, ma andiamolo a dire a chi vive invece nelle aree remote oppure a quanti dovranno chiudere i battenti della propria azienda, perché con questa zona economica speciale (ZES) unica che avete tanto voluto di fatto verranno tagliati dal mercato migliaia di imprenditori delle aree più remote.

oltre che arginare le criticità. Di certo non basterà istituire la Giornata mondiale del *made in Italy*, che cade il 15 aprile di ogni anno, ad evocare il genio italiano per eccellenza, Leonardo da Vinci. Non vorrei qui ricordare il *flop* dell'utilizzo della Venere di Botticelli con «Open to meraviglia» *(Applausi)*, anche perché alla fine le nostre eccellenze verranno poi ad esaurirsi.

di cui si sta parlando in questi tempi, perché di certo è più importante che lo studente venga preparato con una formazione post-diploma, che è quello che manca alle aziende.

nazionali e il tessuto economico industriale del Paese, ma ancora una volta, signor Presidente, le risorse messe a disposizione sono esigue, ridicole e, tra l'altro, spostate sempre da un capitolo all'altro. Il risultato complessivo è un miscuglio di provvedimenti, tutti mancanti di sostanza e soprattutto di dotazione economica, senza considerare che in questo provvedimento non abbiamo letto un solo comma capace di affrontare seriamente la problematica della contraffazione e dell'aggressione alla nostra ossatura produttiva.

Però, come ormai accade puntualmente con ogni provvedimento, questo Governo preferisce una *delivery* mediocre, del tutto irrilevante, piuttosto che ammettere che il film della propaganda, che puntualmente andate proiettando, non fa altro che portare l'Italia, e soprattutto il *made in Italy*, a sbattere contro il fallimento. *(Applausi)*. Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare un provvedimento che, come quello di ieri, ha un titolo molto altisonante ed è molto importante, ma purtroppo, proprio in modo simile a quello che abbiamo visto ieri sul Piano Mattei, anch'esso in realtà è una scatola vuota, nonostante il fatto che avrebbe dovuto assistere una delle colonne, forse la principale, dell'economia italiana. Le nostre esportazioni hanno retto questo Paese durante tutte le grandi crisi economiche che abbiamo avuto dalla fine del secolo scorso ad oggi. L'avanzo della nostra bilancia commerciale, che si è aggirato sempre intorno ai 50 miliardi di euro, ha equivalso ogni anno a una - o due, direi - leggi di bilancio, leggi di bilancio, grazie all'abilità nostra e dei nostri imprenditori di creare prodotti che sono per loro natura destinati al mondo. Gli imprenditori italiani non producono per il mercato domestico, ma fanno cose che, per la loro qualità e la loro capacità di attrarre il cliente globale, sono destinate al mondo. Ovunque ci sia una classe media, lì c'è una richiesta di Italia. Il nostro *made in Italy*, che si è voluto addirittura inserire nel nome del Ministero con una scelta, secondo me, abbastanza opinabile, è comunque certamente una delle nostre colonne.

dei punti di forza e dei punti di debolezza delle nostre aziende esportatrici - che hanno attraversato anche le crisi

Le nostre imprese esportatrici invece sono fortissimamente vocate alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.

un grande "volemose bene" che secondo me non risponde alle grandi crisi di questi tempi. Pensiamo al Covid, all'interruzione delle catene globali del valore o all'aumento dei costi dell'energia, tutte vicende che hanno modificato - direi, anzi, rivoluzionato - il sistema del commercio internazionale in questi anni. Allora, guardando a questo provvedimento, mi vengono alcune riflessioni. Per esempio, sappiamo che il nostro tessuto produttivo è fatto soprattutto da piccole e medie imprese e che per una piccola e media impresa rivolgersi al mercato mondiale è più difficile. Le grandi imprese hanno per loro natura più facilità a esplorare opportunità all'estero. Con i Governi Renzi e Gentiloni - e con il ministro Calenda

con i quali più commerciamo. Trovare un prodotto italiano a New York o sulla West Coast è facile, ma se si abita nel Midwest e si vuole trovare il Parmigiano reggiano è molto probabile che non lo si trovi, quindi bisogna far arrivare lì quei prodotti. Lo si fa? No.

un lavoro in questa direzione. Addirittura si tagliano i fondi per le *startup*, che sono aziende che dovrebbero essere molto sostenute dallo Stato perché hanno una fortissima mortalità in quanto prevedono un grande rischio. Si è tagliato anche il fondo per l'innovazione per creare questo fondo sovrano

vendere in mercati dove oggi ci sono dazi e che domani non ci saranno più. Che fine ha fatto il trattato con il Mercosur? Perché il trattato di libero scambio con l'Australia passa delle giornate pessime? Voi nell'Unione europea con il commissario al commercio state spingendo perché l'Italia e l'Unione europea abbiano trattati di libero scambio sempre più efficienti? Soprattutto, perché non ratificate il CETA, che tutti sappiamo quanto abbia aiutato le aziende italiane ad esportare di più in Canada? Che cosa aspettate? inoltre: quante missioni di sistema avete fatto? Quante volte avete accompagnato le nostre imprese all'estero, soprattutto dove non c'è un'economia di mercato e l'economia è pianificata, quindi essere accompagnati dal proprio Governo è importantissimo per poter piazzare i propri prodotti? State a Roma o andate in giro ad accompagnare le imprese italiane? E le nostre fiere?

praticamente simile ai nostri istituti di ragioneria, tecnici commerciali con una spruzzatina di qualcosa. Ma lo diceva già il collega che parlava prima di me: gli ITS dove sono finiti? Perché non si guarda all'istruzione superiore? Che fine hanno fatto filiere come quella della moda, per esempio? C'è qualcosa sul tessile, ma la moda che è un settore fondamentale delle nostre esportazioni, anche in termini di immagine, dov'è?

un nome attraente dal punto di vista del *marketing* a questo Ministero. Vi dico la verità: se l'aveste chiamato Ministero dello sviluppo economico, come si è sempre chiamato (perché è quello il suo lavoro, ossia sviluppare l'economia del Paese), e se faceste leggi che servono a sviluppare l'economia del Paese, ne saremmo contentissimi. La verità è che da questo questo provvedimento si capisce perfettamente che un'idea di cosa sia il *made in Italy*, di cosa siano le nostre esportazioni e di cosa serva alle nostre imprese esportatrici è lontanissima dall'essere nelle conoscenze di questo Governo. È un'occasione perduta e davvero dispiace, proprio perché sappiamo quanto sia importante, per la nostra economia, poter esportare bene.

Quello che doveva essere la punta di diamante delle disposizioni per valorizzare e promuovere le produzioni identitarie, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali dell'economia del Paese, si è rivelato un altro buco nell'acqua. Ancora una volta, purtroppo, il sistema imprenditoriale delle eccellenze italiane si trova con le ruote sgonfie, davanti a una lunga strada da percorrere, pagine e pagine piene di norme che hanno il solo effetto di uno squillo di tromba. Tutti attenti, ma non segue nessuna azione concreta per il Paese Italia. *(Applausi)*. Ecco dunque che vengono proposte, com'è stato più volte ripetuto, l'istituzione della giornata del *made in Italy*: ne avevamo bisogno; l'introduzione della Fondazione impresa e competenze per il *made in Italy*: ne avevamo bisogno; la costituzione di un ennesimo albo, quello sulle imprese culturali e creative: ne avevamo bisogno; la registrazione dei marchi per i luoghi di cultura: bene, ne saranno felici. Sono tutte iniziative che hanno l'effetto invece di burocratizzare e, ancor peggio, in alcuni casi, di foraggiare architetture normative pedanti inutili: quindi, soldi spesi non si sa per cosa. I contenuti, tra l'altro, stridono fortemente con l'atto d'indirizzo che definisce le priorità politiche del Dicastero delle imprese del *made in Italy* per il 2023. Tra i sei punti prioritari, infatti, il quarto posto è occupato dal concetto di rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese. un concetto che, usando una formula elegante, possiamo dire non sia stato correttamente recepito e probabilmente a questo punto non compreso da chi ha stilato il pacchetto di disposizioni di questo disegno di legge, per di più lasciato fermo per oltre sei mesi. Sorge il dubbio che non fosse chiaro cosa veramente si volesse fare. Si ha l'impressione che si scelga il titolo del provvedimento, purché sia altisonante, e poi lo si riempia in tutta fretta e troppo spesso, purtroppo, se non si fanno danni, si appesantisce il quadro normativo, creando fardelli e quindi caos. È passato un tempo eterno da quando il testo è stato presentato alla Camera, il 27 luglio, se si pensa alla trattazione lampo inferta, invece, a questo ramo del Parlamento, che ha la sola colpa di vedere arrivare questo provvedimento in seconda lettura. Allora, ho un suggerimento per questo Governo. Chiediamo a Babbo Natale un bell'orologio, così da rendervi consapevoli, con le lancette in mano, che non possono passare mesi per l'esame di un testo alla Camera e l'equivalente di una manciata di secondi qui in Senato. *(Applausi)*. Ce lo siamo visto passare davanti

Cosa inversa sta succedendo per la legge di bilancio, con l'aggravio dell'affermazione del presidente Meloni, che il 28 ottobre scorso aveva ribadito di confidare nell'approvazione in tempi brevi. Invece, siamo ancora qui a parlarne. Il 16 ottobre sempre la nostra *Premier* - o il nostro *Premier* - si beava del fatto che la legge di bilancio fosse stata approvata in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'unità di vedute del Consiglio dei ministri e della maggioranza che sostiene il Governo; unità di vedute che, loro malgrado, si è sciolta come neve al sole, anche perché il suono delle parole è esercizio provvisorio, ha fatto tremare le carte su diverse scrivanie negli ultimi giorni e dunque di corsa siamo arrivati a concretizzare. È evidente che tener fede agli impegni presi e ai proclami sulle tempistiche di approvazione è una delle tante cose che non sta riuscendo affatto a questo Esecutivo. Veniamo dunque alla nostra trattazione del disegno di legge in Senato. Le audizioni sono state escluse, sin dalla prima seduta in sede referente, sulla base del fatto che la X Commissione alla Camera aveva svolto un'indagine conoscitiva sul *made in Italy*, approvando un documento conclusivo. Quindi noi, in 9a Commissione qui in Senato, non abbiamo avuto neppure le audizioni. Peccato che questo documento conclusivo, approntato alla Camera, contenesse l'auspicio di semplificazioni delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa e di *export*, oltre che semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *made in Italy* nel commercio con Chi mi ha preceduto ha sottolineato questo aspetto fondamentale per il quale non si è fatto nulla.

ci sono delle semplificazioni. Vi è poi la semplificazione per la filiera della nautica, in particolare le autodichiarazioni sul possesso dei natanti da diporto, anche quelli che navigano su acque straniere; ne saranno felici coloro che possiedono delle imbarcazioni, certamente non i cittadini del ceto medio. Si tratta di questioni che - lo possiamo dire apertamente - non sono centrali nel dare nuova linfa al tessuto economico del settore dell'imprenditoria nazionale. Ancora, vi è l'articolo "Frankenstein" sul liceo del *made in Italy*, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera e che, nel vano tentativo di accordare le varie voci, ha sortito l'effetto di non accontentare nessuno. nessuno. Credo poi che nessuno avvertisse l'esigenza di istituire un marchio per i luoghi della cultura, brandizzando e mercificando i parchi archeologici, i complessi monumentali, i musei, le biblioteche e gli archivi. La conoscenza del patrimonio culturale non si incrementa trattando le nostre bellezze come fossero oggetti a cui infliggere una tacca. I simboli dei luoghi e delle bellezze nazionali hanno una dignità che non può essere calpestata da una mercificazione totalmente fuori luogo. La nostra cultura non ha bisogno di marchi; per creare valore, quindi, l'ultima cosa da fare è proprio introdurre marchi inutili. I *report* sul settore turistico in questo senso parlano chiaro: bisogna far sì che le persone vadano a visitare i posti della cultura, perché calamitate dal fattore attrattivo e soprattutto che tornino in quei luoghi. Bisogna offrire i servizi, la viabilità e tutto ciò che facilita la vita del turista facilita la vita del turista e lo motiva a tornare sui nostri territori. Solo in questo modo si pongono le basi per dar vita a una ricchezza circolare, tesa a massimizzare il coinvolgimento e il pregio, prima di tutto umano, che il nostro patrimonio custodisce. I nostri interventi, quindi, hanno avuto tutti una forte coerenza e un importante obiettivo: dare effettivo risalto al cuore pulsante del sistema imprenditoriale italiano, a partire da quello agroalimentare. La campagna olivicolo-olearia quest'anno a gran voce richiede risposte immediate per quello che è un concreto settore trainante per una filiera turistica davvero *made in Italy*. Per questo abbiamo predisposto un pacchetto a sostegno del settore olivicolo, dalla dalla coltivazione alla tavola, con una difesa a 360 gradi; un rinvigorimento dei controlli anticontraffazione indispensabili per garantire qualità e alimentare la fiducia del consumatore, che davvero può constatare la differenza nel marasma dei prodotti in commercio e, nello stesso tempo, il potenziamento dell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'andamento dei prezzi in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'introduzione di un contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità, a favore delle micro, piccole e medie imprese agricole in forma singola e associata, nonché delle cooperative sociali del settore che realizzano olio EVO 100 per cento italiano: vale a dire un olio le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano. Un altro prodotto agroalimentare caratterizzante è quello del pane ed è per questo che abbiamo proposto l'istituzione di un fondo per sostenerne la produzione, a beneficio delle aziende che usano esclusivamente ingredienti di origine italiana (pensiamo al nostro grano italiano). Abbiamo puntato anche a un incremento del fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura e di quello sul sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Abbiamo spinto per la creazione di nuovi fondi tesi a trainare dei comparti in crescita, fortemente legati alle attuali esigenze di economia circolare e di sostenibilità, come quello della mobilità lenta agro-rurale e quello sugli allevamenti sostenibili. Ma la fretta di una maggioranza dedita solo a fare il pugno duro, visti i suoi numeri, ha impedito che su questi argomenti si potesse innescare una discussione seria e produttiva. Ovviamente tutto il nostro lavoro emendativo è stato rigettato. Amen.

Signor Presidente, il *made in Italy* è ormai un marchio proprio del nostro Paese, che ne identifica non solo i prodotti di eccellenza, ma in un certo qual modo anche lo stile di vita. Il *made in Italy* è quel complesso di sfumature che rende il nostro Paese così amato, imitato e visitato. Che si pensi ad un'azione che possa rafforzare il *made in Italy* in maniera strategica mi sembra un atto opportuno, quanto doveroso. Come opportuno e doveroso sarebbe stato permettere al Senato, in Commissione e in Aula, di discutere nel merito di questo provvedimento e di apportarvi miglioramenti. Invece, ancora una volta, la maggioranza ci propone una procedura monocamerale: un provvedimento così importante, che tratta di questioni che stanno alla base dell'*export*, la maggiore ricchezza del nostro Paese, e che indubbiamente si presterebbe a essere migliorato da una riflessione comune e pacata di tutto il Parlamento, nonché da un potenziale consenso unanime, arriva blindato in seconda lettura al Senato. Non c'è possibilità di migliorarlo e purtroppo questa non è una novità. Se invece ce ne fosse stata data l'opportunità, signor Presidente, avremmo potuto ragionare insieme su quelli che riteniamo essere i quattro punti fondamentali di una legge definita *made in Italy*. punti sono: proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi; fare in modo che questi arrivino all'estero; valorizzare le risorse per la promozione; incoraggiare gli investimenti in Italia. Per quanto riguarda il primo punto (proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi), chiedo ai colleghi di maggioranza - tramite lei, signor Presidente - di ammettere che la tanto vituperata Europa ci ha dato una mano, approvando recentemente, anche grazie all'impegno degli europarlamentari italiani del Partito Democratico, la legge che prevede l'indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. Per noi che vediamo nelle nostre produzioni locali l'eccellenza del *made in Italy*, questa regola rende di per sé praticamente inimitabili i nostri marchi e garantisce l'italianità di ciò che arriva sulle tavole del mondo. Noi siamo favorevoli, senza ombra di dubbio, alle iniziative che salvaguardano il *made in Italy* anche in materia di lavorazione e processi produttivi di qualità. Ma questo provvedimento presenta lacune straordinarie. E qui vengo al secondo punto delle priorità: fare in modo che i prodotti *made in Italy* arrivino all'estero. Abbiamo bisogno di allargare i nostri mercati, per far sì che i prodotti *made in Italy*, ma anche i servizi e il nostro *know-how*, arrivino nei mercati esteri per poter crescere. Il provvedimento in esame però... *(Brusio)*. Presidente, la prego di

Il provvedimento in esame manca però di una visione fondamentale che avrebbe dovuto essere centrale. Mancano la percezione, la funzione e le potenzialità che l'estero ha per il *made in Italy*, che le nostre comunità nel mondo hanno per il *made in Italy*. Serviva una strategia di medio e lungo termine che questo provvedimento, con l'aiuto del Parlamento, avrebbe potuto prevedere per evitare in primo luogo che si facesse confusione;

Ci aspettavamo ad esempio che si affrontasse la questione di come accompagnare le piccole e medie imprese, cioè l'ossatura della nostra economia, la parte più genuina del nostro *made in Italy*, verso l'obiettivo di raggiungere mercati esteri che, ad oggi, per loro sono proibitivi o sembrano tali. Se avessimo avuto l'opportunità di discutere e modificare questo provvedimento, avremmo potuto studiare soluzioni su come fare ad aprire nuove strade o fornire maggiore sostegno a queste aziende, magari utilizzando risorse che già esistono, come le camere di commercio italiane nel mondo. Avremmo potuto parlare delle opzioni possibili per espandere i mercati esteri e forse saremmo riusciti a convincere il Governo e la maggioranza che insegnamento e promozione della lingua e della cultura italiana sono un momento fondamentale del *made in Italy*; sono quegli anelli che congiungono il nostro Paese con mondi differenti ancor prima che lì arrivino i nostri prodotti. Lingua e cultura sono i due elementi essenziali alla base della chimica del *made in Italy* e del suo apprezzamento mondiale. Proprio ieri in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno a mia prima firma, sottoscritto dai colleghi del Partito Democratico Franceschelli e Martella, che impegna il Governo ad aumentare per il prossimo triennio i fondi riservati agli enti gestori di corsi di lingua e cultura all'estero. Questa, signor Presidente, è la prova che anche la maggioranza - forse, io lo spero - ha capito alcuni degli errori e delle miopie di questo provvedimento che addirittura prevede che la giornata del *made in Italy* sia celebrata in Italia, non all'estero. Anche qui abbiamo cercato di rimediare in qualche modo a questa assoluta mancanza di coerenza con l'approvazione in Commissione di un altro ordine del giorno, sempre sottoscritto dai commissari del Partito Democratico, in cui si chiede al Governo di impegnare anche la rete consolare, il sistema Paese e le camere di commercio italiane nel mondo nelle attività che celebrano questa ricorrenza. Alle nostre aziende, ai nostri produttori, ai nostri possibili clienti non serve una giornata nazionalista del *made in Italy*, ma una giornata nazionale che rivolga il suo sguardo al mondo *(Applausi)*, che sia sul palcoscenico del mondo, come come d'altronde avviene per altre ricorrenze simili, come la giornata mondiale della cucina italiana, la settimana della lingua, la giornata del *design*. Tutto considerato però quelli di ieri sono un piccolo passo nella direzione giusta. Si tratta di atti di indirizzo che, se fossero stati inclusi nel provvedimento, avrebbero rappresentato un miglioramento significativo della normativa. Restando in tema di miopie, in questo provvedimento, signor Presidente, ci si è scordati dei sei milioni di cittadini italiani che vivono al di là dei nostri confini nazionali e dei circa 80 milioni di persone di discendenza italiana. Si tratta di imprenditori, artisti, politici, rappresentanti delle istituzioni e della cultura, a cui non bisogna spiegare nulla su cosa sia il *made in Italy* perché non solo lo conoscono bene, ma contribuiscono anche a promuoverlo più di ogni altra legge o azione di *marketing* che si possa strutturare. Nei mercati rionali di Sydney, Melbourne e Brisbane, luoghi che conosco bene, c'è una miriade di giovani artigiani italiani, emigranti di nuovissima generazione che vendono il *made in Italy*: prodotti della loro terra d'origine, *street food*, artigianato e arte a turisti e locali. Non solo: c'è chi si impegna nella sua professione ed eccelle nel segno dell'italianità. Le faccio un esempio simbolico: nella lista dei migliori 50 bar nel mondo, nei primi 15 ne figurano solo due italiani, che si trovano uno a Barcellona e l'altro a Sydney. Entrambi sono locali aperti da giovani emigranti italiani, quegli stessi a cui, fra l'altro, con la scelta scellerata di cambiare le regole dei benefici fiscali per i rimpatriati, questo Governo sta chiudendo la porta in faccia a un possibile ritorno in Italia. Eppure, se il *made in Italy* è un'eccellenza, lo dobbiamo anche a loro. Il provvedimento in esame, signor Presidente, non tiene conto del fatto che sono questi imprenditori, questi professionisti, questi ricercatori e tanti altri che di fatto trasformano il *made in Italy* da parole, da marchio, a parte integrante della vita quotidiana di altri popoli. Sono loro che aprono le porte a nuovi mercati o nuovi prodotti e di questo bisognava tenere conto nel provvedimento in esame e nelle strategie del sistema Paese all'estero.

Dispiace però aver perso un'occasione importante di confronto, nella quale si sarebbe anche potuto parlare più approfonditamente del ruolo che possono giocare le camere di commercio, gli enti gestori che promuovono la cultura e l'insegnamento della lingua italiana, i Comitati degli italiani all'estero e sociali italiane nel mondo. Questa opportunità, signor Presidente, poteva essere sfruttata meglio anche per riuscire nell'intento di attrarre capitali esteri in Italia, utilizzando l'appetibilità del *made in Italy,* che è fatto - lo ripeto - anche di tecnologia, servizi e professionalità altamente qualificate, che possono essere insegnate rafforzando un settore, quello della formazione, che, oltre oltre che implementare al proprio interno, l'Italia può anche esportare, vista l'esigenza mondiale di professionalità altamente qualificate. In conclusione, signor Presidente, c'era tanto su cui discutere, ancor di più da programmare. Eppure, il Governo ha deciso di nuovo di fare da solo, relegando non solo noi dell'opposizione, ma anche i suoi parlamentari di maggioranza, ad un ruolo marginale. Il risultato è che a perderci sono l'Italia e gli italiani di tutto il mondo.

dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

una coltivazione molto utile anche per il ricambio dei terreni, ma soprattutto perché le fibre vengono già utilizzate. Assumere un impegno sulla macchina di trasformazione della canapa diventa importante per l'utilizzo industriale e per le fibre.

parere favorevole, previa riformulazione del secondo impegno come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di introdurre, dopo il primo biennio di avvio del nuovo percorso liceale, eventuali aggiornamenti delle attività formative, di cui

parere contrario su tutti gli emendamenti.

parere favorevole con la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, la accetto. Mi permetto semplicemente di aggiungere che questo ordine del giorno fa seguito a un'interrogazione, svolta in Aula,

ai Comuni per valorizzare e mantenere gli ambienti in montagna, ma diamoli anche agli allevatori che presidiano il territorio. *(Applausi)*.

il mio ordine del giorno era rivolto a comprendere se si trattasse di una questione interpretativa o se effettivamente l'articolo volesse escludere dalle previsioni del Fondo quegli interventi sul paesaggio agricolo e rurale che non ricomprendessero i percorsi degli animali. bene culturale e tradizionale del paesaggio agricolo e rurale ricomprende anche zone in cui ci sono dei percorsi che non sono collegati al passaggio degli animali e sarebbe un peccato non dare la possibilità anche a questo tipo di territorio di usufruire del Fondo al fine di valorizzare questa peculiarità. Diversamente, si rischierebbe di perdere proprio quella tradizione agricola rurale, perché non ci sono i soldi per mantenerla. Penso, per esempio, che in Pianura padana ci sono grandi distese agricole che derivano dal Medioevo, quindi dalla gestione clericale delle abbazie e si creano tanti passaggi tra gli antichi cascinali lombardi e le varie abbazie che sono percorsi bellissimi e che, in questo caso, verrebbero esclusi. Mi sembra un peccato. Insisto pertanto con la relatrice e con il Governo

Signor Presidente, le parole «*made in Italy*» evocano da sempre l'idea di unicità, autenticità, artigianalità, ingegno, orgoglio italiano, l'idea di maestria e di maestranza, la capacità di tramandare e non disperdere le tradizioni, la capacità di innovare e di spostare le sfide sempre un po' più in là, di fare impresa, di

persone, con tutto il suo portato di cultura, dinamiche sociali, tradizioni e capacità di innovare, perché il *made in Italy* non è soltanto un modo di fare, ma soprattutto un modo di essere. Lasciatemi dire che è la cifra del Governo Meloni. Il *made in Italy* è un marchio riconosciuto in tutto il mondo, al pari del patrimonio culturale e artistico italiano. Il *made in Italy* identifica le eccellenze italiane nel campo culturale, enogastronomico, del *design*, dell'architettura, del lusso, dell'imprenditoria. Il *made in Italy* è un segno distintivo esclusivo del nostro Paese; è un segno universalmente riconosciuto di bellezza e qualità; un patrimonio, anche in termini reputazionali, costruito nei secoli grazie anche all'impegno e al lavoro costante e creativo degli italiani in ogni settore. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, compra una parte dell'Italia, una realtà universalmente conosciuta e riconosciuta, al punto che il *made in Italy* è tra i primi tre marchi al mondo come notorietà. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, in altre parole si affida all'eccellenza e alla qualità in termini di assoluta bellezza, *design* e creatività. Tutelare il *made in Italy* e il *made by Italy and italians*, cioè tutelare gli italiani e gli interessi italiani, è da sempre uno dei pilastri e uno dei fondamenti del centrodestra e di questo Governo. Per noi significa andare incontro alle esigenze del mondo produttivo nel suo complesso, industria, impresa e artigianato insieme, per sostenere un patrimonio universalmente riconosciuto inimitabile - e di questo dobbiamo andare orgogliosi. Vogliamo farlo ancor più oggi, senza oneri eccessivi per le casse dello Stato o, peggio, con contributi a pioggia, a dimostrazione che le nostre filiere sanno camminare da sole se adeguatamente sostenute e dotate di nuove risorse, nuove competenze Per questo vogliamo rendere onore alle tante eccellenze che in questo Paese quotidianamente ci rendono orgogliosi di essere italiani e di esportare l'italianità nel resto del mondo. Se infatti fino ad ora l'Italia, a causa di politiche di sviluppo commerciale deboli o miopi, è stata costretta a muoversi al traino degli altri Paesi, merita di prendere la direzione opposta. I nostri prodotti, la nostra creatività e le nostre competenze devono avere il posto che meritano a livello globale. Con questo provvedimento articolato di politica industriale, fortemente voluto dal nostro *Premier*, abbiamo l'obiettivo ambizioso di rimediare i problemi che da sempre gravano sul nostro sistema produttivo: la burocrazia, la lunghezza dei processi amministrativi e giudiziari, la logistica, il dimensionamento delle imprese per aumentarne il valore. Altrettanto ambizioso è il piano di valorizzare e promuovere, in Italia come all'estero, le nostre eccellenze, le nostre radici, la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, fattori da preservare e rafforzare, non solo per tutelare la nostra identità, ma anche per promuovere la crescita dell'economia nazionale, affinché tutto il sistema Paese possa stare al passo con i cambiamenti e le sfide globali. A questo obiettivo rispondono, ad esempio, lo stanziamento, già da quest'anno, di una prima *tranche* di 700 milioni su un miliardo per il nuovo fondo sovrano nazionale, partecipato dal MEF ed aperto anche ad altri fondi privati, che investirà nelle filiere strategiche fin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime. Il fondo sovrano avrà anche il compito di sostenere l'imprenditorialità femminile in agricoltura, tutelare la biodiversità e promuovere i prodotti tipici italiani. È questo il cuore e il motore finanziario del provvedimento. Ma vi sono anche, per esempio, nuovi strumenti per combattere la contraffazione dei prodotti e strumenti per tutelare i *brand* storici in crisi, come il subentro del Mimit, al fine di salvaguardare la continuità. Questo vuol dire tutelare la storia e la cultura del nostro Paese e non solo gli *asset* economici. La formazione, lo sappiamo, resta uno dei tasselli fondamentali quando si parla di crescita e di innovazione. La formazione è la fabbrica del futuro per tutti noi. Il tema dei giovani e dell'occupazione femminile è anche centrale in questo provvedimento. Ecco perché accogliamo con favore l'istituzione, prevista dal disegno di legge, del liceo del *made in Italy*, implementato con l'insegnamento delle discipline STEM: permetterà alle imprese del settore di trovare i professionisti che cercano, in grado di seguire l'innovazione, di stare e competere sul mercato italiano ed estero. Siamo gravemente in ritardo e ci doveva pensare il Governo Meloni. Ci sono poi molte altre misure in questo disegno di legge: l'incentivazione per le *startup*, i *voucher* per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento dei brevetti, il sostegno per l'imprenditoria femminile con 15 milioni di euro, la valorizzazione e la tutela del patrimonio immateriale, il contrasto alla contraffazione e al fenomeno dell'*italian sounding*, che ha un volume di affari stimato in 100 miliardi l'anno che vengono sottratti al nostro Paese mediante l'introduzione di moderni sistemi di etichettatura e di tracciatura. Ancora, misure per la tutela e lo sviluppo del sistema agroalimentare per la diffusione della cultura agroalimentare italiana nel mondo e poi misure per le singole filiere, come quelle della ceramica, del legno, del settore termale e del turismo, della cultura, dello spettacolo e della moda, rispetto alla quale ci si è preoccupati della necessità

produttivi che storicamente caratterizzano i nostri territori. Diciamolo pure, signor Presidente, l'Italia ha ali più grandi del nido in cui l'hanno confinata anni di recessione politica. Noi dobbiamo tornare ad essere più orgogliosi del nostro Paese. Se andiamo all'estero, il sistema Italia è stimatissimo. Recuperiamo, dunque, la nostra autostima. Noi abbiamo delle eccellenze che, se veicolate in un sistema, con una visione progettuale a medio e lungo termine, non sono seconde a nessuno. Possiamo essere i primi al mondo e ce lo meritiamo. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio che il nostro Gruppo Gruppo voterà convintamente a favore di un provvedimento che getta le basi perché il nostro Paese possa tornare a crescere e a dispiegare tutte le proprie potenzialità sui mercati esteri. Un Paese che torna a volare sempre più in alto, come ci insegna proprio chi quotidianamente, grazie al suo impegno e alla propria passione, da sempre scrive quelle belle pagine dell'antica dell'antica e nobile tradizione italiana del saper fare e fare bene. È un orgoglio italiano cui diamo il nostro stimato bentornato, come abbiamo detto alla manifestazione

Vice Ministro, ma come mai lei è qui quest'oggi? Bisogna sapere, infatti, che in questo Governo la competenza sulle esportazioni non appartiene al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si chiama *made in Italy*, ma già dal Governo Conte II la vera competenza sulle nostre esportazioni sta in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero che, per esempio, imprese italiane (ICE), che è diretta da un diplomatico, non a caso. Fu fatta la scelta, col Governo Conte II, di spostare la competenza al Ministero degli affari Questa volta c'è un Ministero del *made in Italy*, ma gli imprenditori non sanno se devono parlare più con gli Esteri, o se devono parlare con l'ex Mise: c'è una grande confusione. Quando il Governo non riesce a dare chiarezza ai suoi interlocutori, che sono le imprese, abbiamo già un grande problema di metodo. Qui c'è un grande assente, il ministro Tajani, già ieri sfiduciato sul piano Mattei, adesso forse sfiduciato anche sulle esportazioni: interessante. Dirò subito che noi ci aspettavamo un

commerciale. Noi abbiamo sempre portato a casa annualmente tra i 40 e i 60 miliardi, che sono multipli di una legge di bilancio; le nostre imprese, che hanno fatto sempre dell'Italia uno dei primi dieci esportatori al mondo, hanno resistito a ogni difficoltà, sono state al passo con gli avanzamenti tecnologici e hanno creato posti di lavoro e valore. Quindi, ci aspettavamo che con la creazione di questo Ministero, sebbene nella confusione delle competenze, sarebbe arrivato un provvedimento davvero strategico, che avrebbe stabilito come aiutare le nostre imprese ad attraversare le grandi difficoltà che ci sono state negli ultimissimi anni: pensiamo al Covid e alla rottura alla rottura delle catene globali del valore; pensiamo alle tensioni sui mercati energetici; pensiamo alle guerre; pensiamo al fatto che con il Covid addirittura il mercato interno è entrato in crisi in qualche momento. Pensavamo che il provvedimento avrebbe affermato, in modo cristallino, una posizione antiprotezionistica di questo Governo, perché il protezionismo è evidentemente il più grande avversario di un Paese come l'Italia. Se noi siamo uno dei dieci più grandi Paesi esportatori al mondo, è evidente che abbiamo bisogno che non esistano dazi e barriere tariffarie, proprio per consentire ai nostri imprenditori di esportare. Dovremmo avere la possibilità di aprire mercati disponibili con un *level playing field*, ossia con pari opportunità,

completamente di vista le esigenze delle nostre imprese. Provo a fare qualche esempio: sappiamo bene che le nostre imprese sono piccole e medie. È evidente che rispetto a Paesi dove le imprese sono molto più grandi delle nostre (non voglio pensare alla Corea, dove ci sono grandissimi conglomerati, ma basti pensare alla Germania) gli investimenti, sia in ricerca e sviluppo, ma anche nel *setup* nel *setup* dell'organizzazione che serve a esportare, sono molto più semplici. Allora, per esempio, avremmo voluto vedere qualche intervento di questo tipo: come aiutare le piccole e medie

dell'*italian sounding*, che certo va protetto anche con dei soldi, però bisogna chiedersi: l'*italian sounding* è soltanto un problema o non è anche un'aspirazione del consumatore globale di acquistare la domanda è: come si fa a portare prodotti italiani nella grande distribuzione in tutto il mondo e a fare in modo che il consumatore che vuole acquistare il prodotto italiano trovi quello autentico e genuino e non sia costretto a comprare l'imitazione, perché magari vive in un Paese ad alta immigrazione italiana? Pensiamo al prosecco in Australia o al *parmesan* negli Stati Uniti. Ebbene, se il consumatore lo trovasse sullo scaffale, probabilmente comprerebbe il prodotto italiano. Cosa fate per aiutare l'arrivo di questi prodotti sugli scaffali? Perché non state finanziando la ricerca e lo sviluppo? Perché vi dimenticate che le nostre esportazioni sono tecnologicamente sempre avanzatissime, anche nei settori tradizionali. Dalla lettura di questo provvedimento veramente sembra un po' l'Italia del mandolino e della pizza, che pure è importantissima e ormai viene prodotta e viene pensata, pensata, come tutto l'agroalimentare, in maniera tecnologicamente avanzata. Cosa si sta facendo in questo caso? Penso a tutto quello che abbiamo fatto, per un'economia manifatturiera come la nostra, con i Governi Renzi e Gentiloni, con Industria 4.0, con il *patent box* e con le norme sulla ricerca e lo sviluppo. Dove sono? E soprattutto, perché avete mollato e lasciato la logica degli incentivi diretti alle imprese e siete tornati sull'idea dei bandi,

invece si vedono ancora un bando, che l'impresa italiana, che spesso fa mecenatismo, ritiene poco utilizzabile. per esempio, al nostro ruolo nel WTO e nell'Unione europea. Stiamo rappresentando posizioni antiprotezionistiche e aperturistiche in quelle sedi? Nell'Unione europea stiamo lavorando per allargare gli accordi di libero scambio, che servono alle nostre imprese a vendere di più? Basti guardare all'esempio del CETA, il trattato con il Canada, che è in esecuzione provvisoria e che l'Italia continua a non ratificare *(Applausi)*, ma non si capisce perché, visto che non soltanto stiamo vendendo di più, ma per la prima volta in Canada le nostre indicazioni geografiche protette vengono protette proprio dal CETA. Prima il Prosciutto di Parma in Canada si doveva vendere come *original prosciutto*, perché Parma era un marchio registrato. Oggi, grazie a quel trattato, possiamo tutelare il Prosciutto di Parma. Allora mi chiedo perché non si facciano accordi con il Mercosur, per esempio, o con l'Australia e con la Nuova Zelanda. L'accordo di libero scambio con il Giappone è stato un successone, ma non richiedeva ratifica. Lavoriamo in quella direzione, per combattere contro i dazi e contro le barriere non tariffarie. Missioni di sistema: vi chiedo davvero di aiutare le nostre imprese a viaggiare e di accompagnarle, come si è fatto al tempo dei Governi Renzi e Gentiloni. Lo fanno i tedeschi e lo fanno i francesi, perché, quando si va in Paesi dove l'economia è pianificata dal Governo, Governo, presentarsi accompagnati dal proprio Governo significa avere un accesso al mercato che altrimenti non si ha. Non si può fare il commercio internazionale soltanto stando seduti a Roma.

Mi sembra che, ancora una volta, qui manchi una visione strategica per settore della nostra economia che è fondamentale e davvero portante. Avete affrontato questa vicenda, che necessiterebbe che necessiterebbe davvero di una visione strategica e complessiva, con un approccio che mira a istituire la Giornata del *made in Italy*. Perché no? Diciamoci la verità, però: se questo è, se si istituisce il liceo del *made in Italy*, invece di insistere sulla formazione formazione degli istituti tecnici superiori, che in Italia mancano, se non c'è un approccio diverso, signor Vice Ministro (e parlo anche ai suoi colleghi della Farnesina, che purtroppo oggi non sono qui in Aula), penso che non faremo

Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche oggi, senza il rispetto dei tempi minimi per svolgere un esame organico e approfondito, ci troviamo a discutere l'ennesimo provvedimento ideologico di questo Governo, un disegno di legge complesso e caotico che, pur sostenendo il sacrosanto bisogno di tutela, promozione e sviluppo delle filiere strategiche nazionali, fiore all'occhiello del nostro Paese in Europa e nel mondo, è disseminato di norme pericolosamente propagandistiche. Nei fatti, più che l'esiguo supporto economico a settori produttivi cruciali per il *made in Italy*, quali il legno, la ceramica e le fibre naturali, la cultura, il turismo e la produzione agroalimentare, in questo provvedimento ciò che si rileva maggiormente è la logica politica dei ricchi premi e *cotillon*, con cui voi della maggioranza siete abituati a distribuire confusamente risorse, gettando fumo negli occhi dei cittadini e delle imprese. Sia ben chiaro: siamo tutti nettamente consapevoli e convinti della necessità di favorire lo sviluppo sostenibile e l'ammodernamento dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, messo a dura prova dalla crisi energetica, dall'inflazione e dagli effetti recessivi del mercato. Siamo però certamente meno sicuri della vostra capacità di gestire questi processi in modo efficace, corretto e soprattutto strutturato, in modo che sia possibile riconoscere una strategia, un metodo, un filo conduttore. Senza un approccio coerente e sistematico, vi siete infatti limitati a fare il classico taglia e cuci, scorporando ingenti risorse da fondi già esistenti. È questa la supernovità, lo spirito innovativo di questo Governo? Avete distribuito risorse a mo' di mancia un po' ovunque, peraltro con buona pace di una programmazione temporale veramente idonea a garantire uno sfruttamento funzionale di tali capitali nel lungo periodo, visto che nel migliore dei casi i finanziamenti per i settori fortunati arrivano solo fino al 2025. È il caso, ad esempio, dell'istituzione del cosiddetto Fondo nazionale del *made in Italy*, per il cui finanziamento del solo anno 2024 sono stati sottratti 300 milioni al *venture capital* costituito a favore delle *startup* e delle piccole e medie imprese innovative. Anche solo questo dato deve far comprendere quanto sia lontana la vostra idea di sviluppo e sostenibilità dalle reali esigenze dei settori produttivi di questo Paese che, nell'ambito di un mercato fortemente globalizzato e sempre più digitalizzato, necessita piuttosto di moderni strumenti che gli consentano di guardare al futuro in un'ottica di ricerca e sviluppo, valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un deciso e necessario ammodernamento e una competitività dei propri comparti produttivi per stare al passo con i tempi e soprattutto con la concorrenza. La vostra preoccupazione di preservare e tramandare le radici culturali nazionali purtroppo si traduce nell'utilizzo di metodi antiquati che di certo non aiutano i nostri comparti produttivi ad affermarsi e consolidarsi sul mercato, a maggior ragione in un contesto internazionale sempre più in evoluzione. È per questo che siamo fortemente preoccupati. fortemente preoccupati. Non basta limitarsi a citare nel provvedimento i principi della sostenibilità ambientale, della transizione energetica e dello sviluppo di un'economia circolare all'interno dei processi produttivi delle filiere della moda e delle fibre tessili per innescare un reale cambio di rotta e raggiungere gli obiettivi europei di neutralità climatica e di decarbonizzazione previsti entro il 2050. Alle parole devono seguire i fatti; servono criteri ambientali per evitare il *greenwashing*, disposizioni normative, misure e strategie da utilizzare affinché la transizione energetica ed ecologica e la digitalizzazione non costituiscano per le imprese solo un onere, ma anche una concreta opportunità di abbattimento dei costi e, di riflesso, di maggiori disponibilità per investimenti e sviluppo sostenibile. Servono incentivi alle aziende per sostenerle nel processo di transizione energetica. Il Governo italiano purtroppo rimane nei binari di un mondo che non esiste più, tanto che le parole e le intenzioni del provvedimento al nostro esame risultano limitate e vuote e suonano come una presa in giro come le note stonate di un *carillon* che continua a incepparsi. Ridicole e vacue sono le norme bandierina che istituiscono la Giornata nazionale del *made in Italy* e il premio annuale di maestro del *made in Italy*, simboli della poca serietà di questo Esecutivo, che baratta la politica dell'impegno e dell'efficacia con quella dell'apparenza. Di questo passo, per tutte le giornate celebrative istituite dal Governo Meloni non basteranno le date presenti nell'anno solare. Dannosa, pericolosa, confusionaria e totalmente inutile per la risoluzione dei problemi che affliggono il nostro sistema scolastico è poi la folle idea di istituire il liceo del *made in Italy,* che di fatto fa sparire i licei economico-sociali. Si parla di 419 scuole statali con non meno di 3.000 classi, senza contare i 116 istituti paritari coinvolti. una decisione propagandistica incomprensibile che, noncurante dei terribili dati che vedono attribuire alla scuola italiana quasi due punti in più della media europea per l'abbandono scolastico precoce, con una forte carenza di strutture scolastiche idonee e una grave mancanza di insegnanti (che, tra parentesi, hanno gli stipendi più bassi in Europa), istituisce un nuovo corso di studi che non si comprende come debba svolgersi, dato che non sono previste ulteriori risorse economiche per il suo sviluppo. una scelta scellerata, che appesantisce le problematiche organizzative già esistenti nel mondo della scuola italiana e subordina la formazione degli studenti unicamente alle esigenze e alle logiche del tessuto socioeconomico, scolorendo l'importante funzione interdisciplinare proveniente dall'apprendimento delle materie umanistiche. La vocazione nazionalista di questo Governo anche nel campo dell'istruzione ci porta indietro di un secolo e ci spaventa non poco. Non da ultimo, è imbarazzante constatare che in questo piano di rivalutazione del settore del *made in Italy* manchi completamente la volontà di attuare un serio programma di valorizzazione e di promozione del comparto turistico, un settore di primo piano nel tessuto economico, sociale e culturale del nostro Paese. Secondo un approccio lesivo e controproducente per l'intera categoria degli operatori turistici e delle imprese che operano nel settore, l'unica misura inserita in questo pannicello caldo del Governo per accrescere l'attrattività dell'Italia, la competitività dell'intero settore turistico e la promozione del patrimonio ricettivo e turistico italiano istituisce un misero comitato nazionale per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica. una misura vergognosa, che non rispetta minimamente le richieste di tutela di coloro che lavorano nel settore, peraltro dannosamente liberalizzato da questo Governo, e che mortifica i veri bisogni del settore turistico attraverso l'inutile istituzione del *manager,* figura che non si sa come possa contribuire alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo. Questo *modus operandi,* conservatore e controproducente, ostacola il progresso a tutti i livelli, impedendo che possano concretamente realizzarsi quelle condizioni attraverso cui promuovere realmente la valorizzazione delle produzioni d'eccellenza e le bellezze storico-artistiche del nostro Paese.

del programma del Governo del centrodestra a cui noi di Forza Italia teniamo di più. Siamo in presenza di un provvedimento molto articolato, sia per il numero delle norme (ben 59 articoli), sia per la specificità dei contenuti. un disegno di legge cui ha lavorato il Parlamento e che, pur essendo d'iniziativa governativa, nasce da un lungo lavoro di confronto con tutti gli *stakeholder,* svolto nell'apposita indagine conoscitiva della Commissione attività produttive, commercio Lo scopo è quello di tutelare e accompagnare le nostre filiere produttive e renderle immediatamente riconoscibili, quindi uniche nel contesto internazionale. Lo scopo è quello di tutelare e far apprezzare al mondo il valore aggiunto della creatività italiana, della competenza italiana, delle lavorazioni italiane e dei prodotti che hanno il marchio di *made in Italy*. un disegno di legge che intendiamo approvare entro la fine dell'anno, affinché le sue misure e le risorse economiche che lo accompagnano, pari a un miliardo di euro, siano immediatamente operative. Dal provvedimento emerge chiaramente la volontà di promuovere all'estero i nostri marchi e anche l'idea che a promuoverli siano le donne e quindi un articolo è dedicato all'imprenditoria femminile e all'impresa a prevalente partecipazione femminile. Alla proprietà industriale viene dato il giusto riconoscimento attraverso norme che incentivano la conoscenza e la consapevolezza dei brevetti, cioè dell'importanza di valorizzare i processi di innovazione e i risultati che spesso sono prodotti unici, che vanno assolutamente tutelati. Troppi sono nel mondo i tentativi di imitazione e di plagio di prodotti italiani, di nomi che hanno un suono che ricorda quello del prodotto unico e originale prodotto in Italia. che gli anglosassoni hanno addirittura un termine, *italian sounding*, per significare appunto tutto ciò che suona un po' italiano. Facciamo degli esempi: il *parmesan*, la *salsa pomarola*, gli *spagheroni*, il perché bisogna tutelare il prodotto italiano e la sua unicità. Il disegno di legge prevede inoltre una serie di misure che tutelano la peculiarità delle filiere produttive italiane. Tra queste, quelle del legno per arredo, dell'olio vergine italiano, del tessile, della nautica, della ceramica, del pane fresco, della pasta e della moda. Viene inoltre istituito il liceo del *made in Italy*, cioè un percorso di studi superiori che dovrà essere regolamentato dal Ministero dell'istruzione e del merito. Viene istituita una fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*, con lo scopo di creare un raccordo tra imprese che rappresentano le eccellenze italiane e gli studenti. studenti. L'idea di valorizzare il merito, che è fondamento di ogni eccellenza italiana, è quindi alla base di queste nuove norme. Viene istituita, inoltre, l'Esposizione permanente del *made in Italy* per promuovere in modo stabile l'eccellenza del prodotto italiano di qualità superiore. Si pensa anche di promuovere sia il patrimonio culturale immateriale sia i luoghi di cultura, ma anche di rafforzare la tutela dei siti Internet che promuovono il patrimonio culturale. Il disegno di legge contiene una serie di misure a tutela della creatività delle imprese impegnate nella creazione e divulgazione di contenuti creativi e della loro promozione nel mondo. Sono presenti disposizioni per promuovere il turismo in Italia anche attraverso il potenziamento degli uffici consolari dei Paesi ad alta intensità di flussi turistici. Altri settori da sostenere sono le fiere e i mercati rionali, che possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione dei prodotti italiani. Un capitolo importante e specifici articoli sono dedicati alla cucina italiana, alla certificazione di qualità della nostra ristorazione e alla sua promozione all'estero, così come vengono protetti ulteriormente i prodotti che hanno una specifica indicazione geografica registrata che certifica la loro produzione in determinate parti d'Italia, il legame di quei sapori con il territorio e la loro unicità, indicata dal fatto che quel marchio è producibile solo in Italia. Con essi, vanno potenziate le pratiche tradizionali, i distretti del prodotto tipico italiano e le associazioni che valorizzano le produzioni agricole di pregio. Una svolta nella protezione del *made in Italy* potrà avvenire con l'approvazione dell'apposito contrassegno, una sorta di *brand* immediatamente riconoscibile, che dovrà contraddistinguere l'origine italiana dei prodotti. Riteniamo profondamente innovativa anche l'idea di tutelare le filiere che producono i prodotti italiani attraverso i registri distribuiti, le cosiddette *blockchain*. Infine, un capitolo è dedicato alla lotta alla contraffazione, con disposizioni che partono dalle modifiche ai codici penale e di procedura penale, per arrivare fino alla specifica formazione che deve avere chi si occupa di questi temi in ambito giudiziario e all'introduzione di nuove sanzioni amministrative. di una serie di norme che sono frutto di un lungo confronto con le categorie, con tutti gli esperti e con gli *stakeholder* che hanno chiesto al Parlamento gli interventi che noi abbiamo fatto nostri, dando loro una logica normativa. Crediamo che queste norme saranno efficaci e segneranno un cambio di passo nel tutelare l'eccellenza nel nostro Paese. Oggi diciamo con forza che quello che è fatto in Italia è fatto bene e va tutelato. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

e la tutela del *made in Italy*. Il nome è altisonante e, come si è visto sotto il profilo della comunicazione politica, anche accattivante, intrigante e suggestivo, direi. Peccato che il Senato della Repubblica non sia un cartellone pubblicitario dove affiggere lo *slogan* o il *tweet* della settimana, ma un ramo di quell'istituzione che dovrebbe lavorare su temi concreti e su proposte reali per cercare di migliorarlo, questo Paese. però che per un Governo che ha imperniato il suo operato quotidiano sull'esautoramento delle funzioni del Parlamento e di tutti noi parlamentari, l'Aula di Palazzo Madama si è trasformata in un megafono propagandistico delle finte politiche, perché di concreto, in quello che è passato qui dentro, c'è veramente poco.

è stata quella di promettere soluzioni immediate a problemi complessi. Quest'anno non avete solo calpestato il Parlamento, compresi i componenti della maggioranza, consapevoli e non, costretti pedissequamente a ritirare gli emendamenti perché o non in linea con le vostre politiche scellerate o, peggio ancora, perché gli uffici del Ministero non sono stati in grado di condurre le adeguate istruttorie alle politiche scellerate di cui sopra. Il lavoro di questo Governo si è sostanziato in continui e costanti *slogan* elettorali, mancando completamente di rispetto a questo Parlamento. Ne sono un esempio la legge di bilancio, l'utilizzo spropositato della fiducia, per di più in maniera costante sui decreti-legge, per non parlare del continuo ricorso a decreti-legge *omnibus*, un *modus operandi* profondamente scorretto nei confronti di quest'Assemblea e di tutti i colleghi, per primi quelli della maggioranza; ma pazienza, l'importante, anzi, è che sui *social media* possiate mettere uno *slogan* e qualche video da trenta secondi per accaparrare tanti *like*. Presidente - potevate chiedere al signor Musk di consigliarvi sulla strategia *digital* da utilizzare e magari potete anche chiedergli cosa ne pensa della GPA o della cannabis legale. Vedete, le vostre contraddizioni politiche, alla fine, saltano sempre fuori. Tentate di nasconderle, di sviare e di richiamare l'attenzione su altro, ma alla fine le vostre mancanze e le vostre negligenze vengono sempre a galla. Riguardo al provvedimento in esame, tralasciando il fatto che la bozza di questo disegno di legge circolava da quasi un anno, sarebbe interessante analizzare le motivazioni che vi hanno condotto ad aspettare la sessione di bilancio, ma anche qui pongo una domanda retorica: la risposta è chiarissima. Intasare il Parlamento significa ridurre la possibilità emendativa, quindi ribadire la vostra logica istituzionale secondo cui il Parlamento è sostanzialmente un passacarte. Sul contenuto del provvedimento vi devo dire, però, che in un primo momento ci siamo anche stupiti della quantità di filiere e di settori interessati. Poi abbiamo iniziato a leggere e lì è cascato il vostro castello di sabbia.

Insomma, più che un provvedimento di sostanza, sembra la lista dei desideri e, in maniera più realistica, la lista dei temi da toccare secondo il piano editoriale della comunicazione. Di sostanza ce n'è poca, pochissima: sono provvedimenti estemporanei, provvisori e parziali, una serie di toppe messe qui e lì per sopperire, da un lato, al fatto che vi siete dimenticati di governare un Paese in crisi e, dall'altro lato, per porre rimedio ad una legge di bilancio inconsistente. Il vostro gioco è chiaro, quello di fare solo comunicazione e propaganda e forse è venuto il momento di mettere sempre in evidenza le vostre contraddizioni in tutti i contesti possibili,

Eppure, tante aziende italiane che fanno *made in Italy* stentano ad arrivare a fine mese o a fine anno. Allora mi sono chiesto: qual è il problema? Credo che ne esista una serie, perché forse negli anni passati chi ha governato non ha fatto quello che doveva; non è uno scaricabarile, perché la responsabilità forse è un po' di tutti.

Penso a un aspetto fiscale, perché oltre a quello che ho detto, vediamo che le rimanenze fiscali in questo Paese, come diceva molto bene il mio collega Massimo Garavaglia, nel 2018 erano di 800 miliardi, mentre sono diventate 1.150 nel 2021 nel 2021 (+350 miliardi). Questo si collega inscindibilmente a quello che una parte politica ha sempre ritenuto dell'impresa: c'è stata un'inversione e non c'è stata più nei confronti dell'imprenditore una presunzione di innocenza, bensì una presunzione di colpevolezza, una presunzione di colpevolezza, che ha portato ad appesantire qualsiasi attività e qualsiasi processo abbia dovuto seguire un imprenditore, appesantendolo inevitabilmente. Ciò è avvenuto perché forse chi ha governato in passato si è preoccupato solo del sondaggio del giorno dopo e della prossima elezione, smettendo di avere una visione:

Difesa del *made in Italy* significa inscindibilmente difesa delle comunità locali, a vantaggio e nell'interesse delle future generazioni.

ai 100 miliardi e si traduce anche in una perdita di miliardi di euro di gettito fiscale per l'Italia; l'istituzione di un liceo del *made in Italy* e anche il potenziamento di una serie di strutture - penso all'ICE, alla Simest o alla SACE - e che potrebbero aiutare le imprese, soprattutto anche le più piccole, in particolare quelle dell'artigianato di alta gamma, che rappresenta l'orgoglio della manifattura italiana e verso il quale questo provvedimento si indirizza per poter essere d'aiuto. Credo dunque che questo sia l'ennesimo provvedimento di un Governo, di una maggioranza e, nello specifico, della Lega che stanno decidendo di pensare all'Italia del 2040 e non solo al prossimo sondaggio. Concludo dicendo una cosa, che sembrerà banale, ma che sfugge spesso ai più:

Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, scegliendo la strada del disegno di legge, il Governo ha rinunciato per una volta a toccare ulteriormente il *record* che gli appartiene in modo indiscusso, cioè quello dell'uso e dell'abuso dei decreti-legge che, da oltre un anno, stanno svilendo e mortificando il ruolo del Parlamento. fa ricorso alla decretazione d'urgenza anche quando di urgenza non c'è traccia, in abbinamento pressoché costante con la richiesta del voto di fiducia da parte di un Governo che si dice politico che dispone di una solida maggioranza. È però evidente - e a questo punto è più di un sospetto - che così solida non è. Aver presentato però un disegno di legge non significa che si sia interrotta la prassi che ha già provocato tanti guasti alla vita parlamentare e alla coerenza con il dettato costituzionale, perché anche l'*iter* di questo provvedimento dimostra quanto ormai siamo dentro un monocameralismo di fatto e alternato, in cui la possibilità di emendare un testo è riservata solo a una delle due Camere. Il mancato rispetto per il Parlamento è testimoniato dall'assoluta ignoranza delle dinamiche parlamentari. Stanziare dei fondi, tra l'altro pochi, per l'anno in corso, chiedendo al secondo ramo del Parlamento un esame veloce, cioè di fare presto, pena la perdita di questi pochi fondi, significa aver già deciso che le Camere non discuteranno non svolgeranno fino in fondo il proprio ruolo, neanche di fronte a un provvedimento non urgente e non legato al PNRR, né ad alcun tipo di scadenza costituzionale, se non quelle legate alla carenza di rispetto verso il Parlamento e verso i legislatori, che siamo appunto noi. Come se non bastasse, ciò a fronte di una legge di bilancio che ha aperto altri sciagurati orizzonti, considerato l'invito-ordine ai colleghi della maggioranza di non presentare emendamenti, come vedremo da qui a poco, anche in quest'Aula, per non disturbare un manovratore che, peraltro, non ha nemmeno una rotta precisa e non sa nemmeno bene in quale direzione andare. Lo dimostra perfettamente il provvedimento che stiamo per votare: l'ennesimo *spot* girato usando una scatola ben incartata, ma sostanzialmente vuota; l'ennesimo articolato puramente narrativo, dopo che un titolo, che sarebbe stato anche suggestivo e che muoverebbe curiosità e interesse, dimostra che, in realtà, non ha alcun interesse per la valorizzazione, la promozione e la tutela del nostro *made in Italy*, che pure sarebbe così importante e che ha attraversato

se ormai conosciamo l'improvvisazione e l'inadeguatezza questo Governo e di questa maggioranza, restiamo delusi, sì, e direi anche preoccupati. Nel momento in cui il Paese sta affrontando una serie di criticità

di una strategia di difesa dei nostri *asset* industriali, delle nostre imprese, del nostro *export* e della nostra competitività nei mercati internazionali. Arriverei a dire che, nel nostro mondo globalizzato, siamo di fronte a delle sfide ineludibili. Pensiamo a quanto accaduto alla COP28, al consenso che la comunità internazionale, pur tra mille difficoltà e resistenze, ha raggiunto sull'abbandono dei combustibili fossili e alla necessità che ora anche l'Italia sappia governare i processi di transizione, per dare un pieno e rapido contributo alla concreta attuazione di quanto deciso. Rispetto a tutto questo, però, nulla. Ci troviamo di fronte a un provvedimento che - come hanno detto altri colleghi, definendolo in vari modi - è solamente una goccia nel mare, con l'aggravante che almeno questa volta le premesse per svolgere un lavoro dignitoso c'erano tutte e c'era il tempo sufficiente per ascoltare pezzi importanti del nostro Paese, le parti sociali delle filiere produttive, quelle che si occupano di creatività e di eccellenza italiana. E c'era anche la piena responsabilità da parte nostra, del Partito Democratico e di tutte le opposizioni, di fare un lavoro a tutela del nostro *made in Italy*, specificando bene che cosa serve al manifatturiero, cosa serve al turismo, cosa serve alla meccanica e alle automobili, cioè tutto ciò che certifica l'importanza del *made in Italy* nel mondo. Tutto questo non si è fatto, le premesse sono state deluse e il risultato è veramente disarmante. Faccio un esempio per tutti: il fondo sovrano, poi frettolosamente ribattezzato Fondo nazionale. Comunque lo si chiami, la realtà è che non è nemmeno lontanamente sufficiente per realizzare lo scopo per cui è stato creato. La sua dotazione è ridicola: 700 milioni per il 2023, 300 milioni per il 2024; un miliardo in tutto, mentre la Germania ne stanzia circa 25, l'Irlanda e la Spagna 15 e anche la Grecia 7,5. Dove volete andare con quei 700 milioni? Non sono nemmeno soldi nuovi in realtà, perché sono stanziamenti previsti da altri fondi quindi, una sorta di partita di giro e vorrei dire anche di presa in giro. Che senso ha istituire un fondo che non è in grado di svolgere questo ruolo sistemico e non ha obiettivi chiari, ma anzi rischia di intralciare altri fondi esistenti? Che dire ancora dell'istituzione del liceo per il *made in Italy*, che non solo appare inutile, ma fa anche confusione, andando a sovrapporsi con percorsi già esistenti che funzionano da anni e indebolendo una di quelle leve principali su cui dobbiamo puntare, cioè quella delle competenze, in particolare di quelle tecniche e scientifiche? Penso agli istituti tecnici superiori, su cui invece registriamo ancora ritardi e differenze di genere territoriali. La verità è che siamo - com'è già avvenuto ieri

per avere qualche bandierina da sventolare, ma i risultati sono veramente scarsi, perché a scorrere bene questi articoli non si trova altro che un elenco infinito di coriandoli, estemporanee e interventi parcellizzati privi di organicità, soprattutto privi di efficacia. Non c'è la minima visione di cosa sono e dove devono andare il nostro manifatturiero, il nostro artigianato di qualità, la nostra filiera agroalimentare. non si indica - cosa di cui ci sarebbe bisogno - che cosa si intende fare per il comparto chimico, per esempio, per reggere la competizione del futuro. Non si indica cosa bisognerebbe fare per la nostra siderurgia per procedere lungo la strada della decarbonizzazione, così come nel campo delle telecomunicazioni, oppure di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale. Su tutto questo ci dovremmo confrontare con il resto del mondo e così non avviene. Possiamo capire quanto sia sia radicata e antica la vostra visione autarchica e quanto questo sia un retaggio culturale della destra. Ma non potete trascinare il Paese nelle sabbie mobili della vostra ideologia e della vostra avversione al futuro. D'altra parte, su tutto ciò che è industria ed economia state dimostrando che così pronti non eravate, a tutela dei lavoratori, di cui non vi interessa nulla. Però confesso che, almeno sul *made in Italy*, almeno sulla promozione dell'Italia all'estero, almeno sulla tutela dei prodotti italiani, ci saremmo aspettati da voi un'idea diversa. Non dico tante idee, ma almeno un'idea. Invece nulla, solo propaganda e demagogia, che finiranno per scontrarsi con la realtà. E, badate: non dovete preoccuparvi solo della nostra opposizione, che continuerà ad essere ferma, intransigente e ad appoggiare i suoi contenuti. Vi deve preoccupare - non so se di questo ve ne rendiate conto - la pessima considerazione che questo provvedimento sta riscuotendo lungo i gangli vitali del Paese che produce e che ogni giorno si confronta con i mercati internazionali. Insomma, avete paura di affrontare i veri nodi. Avete paura di affrontare le crisi industriali. Non avete una strategia. Avete paura di affrontare

colleghe, Vice Ministro, ancora una volta Fratelli d'Italia - si può dire tutto quello che si vuole - e il suo Governo mantengono la parola data ai propri elettori. Nel nostro programma è sempre messa la necessità di promuovere il *made in Italy*, il *brand* Italia, le eccellenze italiane in campo culturale, enogastronomico, del *design*, dell'architettura e dell'imprenditoria tutta. Abbiamo già affrontato la tutela della proprietà intellettuale in un precedente provvedimento. Quello che ci impegna oggi è un ulteriore passo in avanti nella direzione giusta. La forza del *made in Italy* è la *slow production* e la *slow manufacturing*, cioè produrre con i tempi giusti prodotti di grande qualità, rispettando anche la persona e le sue relazioni con la società. Sto parlando di quell'umanesimo industriale che ha inventato Adriano Olivetti, grande imprenditore del nostro Paese *(Applausi)*, purtroppo a volte un po' dimenticato (lo conoscono di più all'estero). Dovremmo davvero fare qualche cosa per riproporre tutto il suo pensiero dell'umanesimo industriale. Il *made in Italy* ci consente di produrre prodotti di qualità, spesso non seriali, perché la differenza della nostra filiera produttiva

Il marchio *made in Italy* - lo abbiamo già detto tutti - è stato decretato da KPMG, una delle *big four*, al terzo posto, dopo Coca-Cola e Visa. Ma questo non vuol dire che la sfida che possiamo affrontare tutti insieme non sia quella di fare un *upgrade*, un *ramp up* di questo marchio e portarlo ancora più in alto. Dobbiamo riuscire tutti insieme a portare la *reputation* del *made in Italy* ancora più in alto, verso

Noi dobbiamo riuscire, perché abbiamo un *made in Italy* nascosto in Italia, quello delle micro-imprese. Le micro-imprese non sono tracciate, ma fanno dei prodotti di grandissima qualità e unici. Queste micro-imprese sono il futuro del nostro Paese, per portare ancora più in alto il *made in Italy*. Una microimpresa non ha la possibilità di fare internazionalizzazione e di fare *marketing* ed è per questo che, con la cabina di regia, noi dobbiamo aiutarla e portarla avanti. Sappiamo tutti che queste imprese hanno dei prodotti straordinari, conosciuti però semplicemente nel loro ambito locale.

che gli italiani sono dei grandissimi e bravi trasformatori; creano dei prodotti trasformando delle materie prime e facendone dei prodotti unici. Questa è la nostra forza, questa la nostra capacità.

investimenti. Questo è il principio della fine; c'è un bellissimo libro che ne spiega le ragioni. Noi dobbiamo avere fame di crescita, gli imprenditori devono avere sempre fame di crescita.

persone. L'imprenditore, se veramente tale, ha una innata propensione a investire in ricerca e sviluppo; per continuare a migliorare se stesso e la propria azienda c'è bisogno che i capitali siano ben vestiti e, dall'altro lato, ci siano delle persone formate formate in grado di sfruttare questa opportunità. Per questo motivo ben venga la politica che sta portando avanti il Ministero dell'istruzione e del merito con la costituzione del liceo del *made in Italy* e lo sviluppo degli ITS. Non è vero che non ci stiamo occupando degli ITS, non è assolutamente vero. Ricordiamoci che solo due anni fa la Germania ne aveva 800 e l'Italia ne aveva 100; oggi ne ha molti di più, sta procedendo in questo percorso. È un tipo di formazione che serve alle aziende ed è quello che stiamo facendo. Ripeto quindi che non è vero che non li stiamo facendo e non li stiamo prendendo in considerazione.

a quel mercato di prodotti che presentano nomi e *slogan* riconducibili al nostro Paese, ma che nulla hanno a che fare con l'Italia, rappresentando invece il mercato del falso italiano con l'intento evocativo del *made in Italy*. Il nostro settore agroalimentare vale 60 miliardi, quello dell'*italian sounding* ne vale quasi il doppio; la produzione italiana è cioè sorpassata dal finto cibo italiano. Per questo motivo, nel confronto tra le imprese,

poi il prosciutto di Parma, il San Daniele, la mortadella di Bologna, l'olio extravergine e le conserve di pomodoro. Da un punto di vista legislativo, non si tratta di prodotti contraffatti, non essendoci violazioni del marchio registrato. Non riusciamo quindi legalmente né a perseguirli né a punirli. Quei prodotti hanno solo una valenza evocativa che ricorda l'italianità del prodotto al fine di indurre il consumatore ad associare erroneamente quei prodotti con il *made in Italy*. I maggiori produttori di tutto questo sappiamo essere in America, in Canada, in Francia e in Germania. Questo fenomeno ha due aspetti negativi fondamentali: colpisce i produttori italiani, sottraendo grosse fette di mercato, e i consumatori che comprano prodotti spesso di bassa qualità, credendo di comprare invece un prodotto di eccellenza. In questo modo si reca anche un danno

crede di comprare prodotti italiani. Quello è il mercato che noi dobbiamo andare a aggredire e a conquistare. C'è bisogno di una riduzione della burocrazia, delle barriere tariffarie e doganali per favorire il commercio dei prodotti *made in Italy* a discapito di quelli falsi. Le nostre istituzioni devono opporsi al fenomeno in modo compatto, portando avanti all'estero politiche di promozione del vero cibo italiano. Bisogna proteggere in modo assoluto il nostro *brand* identificativo, tracciando il prodotto lungo tutta la filiera.

è un soggetto visionario e innovatore che, con impegno, non fa altro che dare corpo a un sogno, assieme ad altre persone che lavorano non per lui, ma con lui. Se c'è crisi, le grandi aziende licenziano, le nuove investono. La parola d'ordine deve essere crescita. Bisogna aumentare la percentuale di occupati, di donne e di laureati, anche con l'aiuto di un'immigrazione di qualità che ci possa dare una mano. Concludo questo intervento, che non credo sia stato polemico, perché ho scoperto che la polemica gli imprenditori non la fanno, avendo scoperto che non la fatturano, per cui è poco attrattiva. *(Applausi)*. Per parafrasare

una sposa bambina che si trovava in carcere da dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per aver ucciso suo marito dopo anni di violenze. È l'ennesima notizia inaccettabile. È stata impiccata dal regime iraniano e dalla sua macchina omicida. Oggi un'altra donna è stata uccisa brutalmente, calpestando la tutela dei diritti umani e confermando l'orrore del regime degli *ayatollah.* tutta la mia vicinanza alle coraggiose donne che si battono in Iran e nel mondo per difendere i loro diritti e la loro libertà. L'Italia e tutti noi siamo al fianco delle donne per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà.

appende per il collo i figli dell'Iran, che spesso combattono per la libertà e per la dignità, e spesso sono donne. L'Iran è il Paese al mondo -

che era stata una sposa bambina ed era stata messa nelle mani di un uomo molto più grande di lei, che l'aveva fatta oggetto di violenze, che l'aveva violentata in senso fisico e morale e che lei aveva ucciso. Ci sono due cose che io penso sia molto importante dire. La prima è che il regime degli *ayatollah* iraniani deve sapere che il mondo li guarda che questa Repubblica e questo Parlamento hanno gli occhi aperti su quello che succede in Iran. Non pensino che tutto questo avvenga lontano dallo sguardo del mondo. Lo dico con precisione alla rappresentanza diplomatica di Teheran qui a Roma e chiedo al ministro degli affari esteri Tajani di farsi portatore di questo messaggio del Senato italiano presso l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran a Roma.

che è la privatizzazione della giustizia penale, perché Samira è stata uccisa questa mattina in quanto la famiglia del marito non ha concesso il perdono. Ricordiamo sempre che anche nel nostro Paese le sentenze penali vengono emesse e vengono pronunciate in nome del popolo italiano. Il diritto penale non è materia privatistica, non serve a dare direttamente soddisfazione alle vittime. Il giudice penale non è l'arbitro tra due contendenti. Le sentenze penali vengono pronunciate in nome del popolo italiano e sempre bisogna ricordare il diritto degli imputati di vedersi riconosciuti innocenti a prova contraria e fino a giudizio definitivo. Non si può pensare che la vita di quella donna sia dipesa dal mancato perdono di un'altra famiglia. È una cosa intollerabile e, insieme all'idea che sia stata uccisa per mano dello Stato, penso sia il doppio della barbarie.

a cui vengono sottratti ogni possibilità, ogni futuro e anche la propria infanzia e i diritti che porta con sé. Questa sposa bambina è stata da un Paese che sta calpestando i diritti umani e - ahimè - devo registrare con una scarsa presa di posizione da parte delle organizzazioni internazionali, a cominciare

di cui sentiamo in questo momento tutto il dolore e certamente l'indignazione per il supplizio a cui quella ragazza è stata sottoposta. Alziamo davvero la voce da qui nei confronti dell'Iran.

è stato già illustrato - è un ex sposa bambina che ha avuto una vita bersagliata da atti di violenza commessi proprio da quell'uomo che poi lei ha ucciso. Questa esecuzione ha scosso l'opinione pubblica italiana, ma direi l'opinione pubblica mondiale. È motivo di grande delusione e di profondo sdegno il fatto che i tanti appelli che si sono succeduti nell'ultimo periodo per la sua salvezza siano caduti nel vuoto. L'Iran, pur non avendo aderito alla moratoria delle esecuzioni promossa dalle Nazioni Unite, ha ratificato comunque atti internazionali importanti che si basano sul rispetto della vita umana. Faccio un appello tramite questa Aula all'ambasciatore dell'Iran in Italia perché, nella sua funzione di rappresentante di uno Stato dalla storia millenaria, possa svolgere un ruolo prezioso affinché l'Iran attivi velocemente il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, a cominciare proprio dal diritto alla vita. *(Applausi)*. Noi, come comunità e come rappresentanti di quest'Assemblea così importante, non possiamo far finta di nulla davanti a questa triste

per la tutela e il rispetto dei diritti umani, inoltrerò una richiesta formale all'ambasciatore. Signor Presidente, a volte il caso sa essere davvero beffardo, in un certo senso. Nelle stesse ore in cui ci è toccato probabilmente tirare un triste sospiro di sollievo, perché abbiamo saputo che i genitori di Saman sono stati condannati all'ergastolo - Saman era una ragazza di origine pakistana destinata ad un matrimonio forzato, la cui ribellione le è costata la morte qui nel nostro Paese - purtroppo abbiamo appreso anche della notizia dell'esecuzione barbarica, sia nel metodo che nel merito, avvenuta ai danni

i figli avuti dal suo aguzzino, quello che la società aveva imposto divenisse suo marito. E non c'è stato nulla da fare, nonostante gli appelli di Amnesty International, di altre organizzazioni non governative e nonostante una certa pressione, probabilmente non sufficiente, come è stato detto anche dagli interventi precedenti, sul regime iraniano. Non sono bastati purtroppo a risparmiarle la pena inflittale. Io sono orgogliosa di far parte del Parlamento che nella scorsa legislatura ha approvato norme più stringenti che contrastano il fenomeno dei matrimoni forzati anche qui nel nostro Paese. Così come sono orgogliosa del fatto che i componenti e il Presidente del Gruppo interparlamentare, intendono sostenere la resistenza in Iran, perché esiste una resistenza in Iran. Quindi io non posso far altro che unirmi agli appelli che sono stati fatti in precedenza anche dalla collega Pucciarelli, perché questo Senato, che da sempre anche nel Paese è riconosciuto come un baluardo per la difesa dei diritti umani non solo in Italia, ma nel mondo, possa davvero farsi sentire e possa far sentire che l'attenzione

la collega Pucciarelli, hanno pronunciato. Vorrei chiedere però alla Presidenza cosa è possibile fare per evitare che questo tema

lo chiedo a lei, come Presidente - a svolgere una riflessione maggiore su questo tema e a dare una continuità non solo a livello di solidarietà - certo, la solidarietà è importante - per far sì che non vi sia solo un messaggio all'ambasciatore. Bisogna che il Parlamento italiano assuma posizioni determinanti e dia un messaggio più forte. In queste occasioni

aveva un bambino nel ventre. Con sette coltellate poche ore fa è stata uccisa, molto probabilmente dal presunto *stalker* che aveva denunciato qualche mese fa. oltre all'Iran, dobbiamo considerare che anche nel nostro Paese succedono ancora cose del genere. Penso che in questo momento il Senato della Repubblica debba stringersi nei confronti della famiglia e soprattutto della comunità di Treviso. *(Applausi)*. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 18,30 con la discussione del disegno di legge di bilancio. *(La

voglio iniziare dalla fase dei ringraziamenti. Innanzitutto, saluto e ringrazio il sottosegretario Savino, ma vorrei ringraziare tutto il Governo, dal ministro Giorgetti al ministro Ciriani, i sottosegretari

gli altri due relatori, i senatori Liris e Damiani, ma soprattutto i componenti della 5a Commissione per il lavoro svolto, anche in maniera ordinata.

È stato un lavoro abbastanza lungo. Abbiamo iniziato con le audizioni nella giornata del 7 novembre e per questo voglio ringraziare anche tutte le parti sociali che sono intervenute a portare il loro contributo e la loro esperienza,

contestualizzato: usciamo dal periodo del dopo Covid, seguito dalla guerra in Ucraina e poi dall'ultimo conflitto che è esploso tra Israele e Palestina.

sull'aiuto a famiglie e lavoratori e gran parte di questa manovra di bilancio si prefigge, appunto, di dare sostegno a famiglie e lavoratori, soprattutto quelle dei redditi medio-bassi. Il disegno di legge di bilancio contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Il disegno di legge è suddiviso in due sezioni, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, ed è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF. Nel merito, la legge di bilancio è suddivisa in titoli: risultati differenziali del bilancio di Stato; misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie;

giustizia; misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina; misure in materia di calamità naturali ed emergenze; enti territoriali; disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali. Partendo da alcuni articoli che ho cercato di sintetizzare, per dare un po' di coscienza anche a chi non ha seguito nel merito i lavori, l'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e di cassa. L'articolo 2 istituisce il fondo per indigenti per acquisto di beni di prima necessità. L'articolo 3 istituisce il fondo di garanzia per la prima casa, esteso anche alle famiglie numerose. L'articolo 4 stanzia 200 milioni per il bonus elettrico. L'articolo 5 reintroduce il taglio del cuneo fiscale, cioè la misura che dicevo prima, che serve per sostenere i lavoratori delle fasce medio-basse. All'articolo 6 vengono introdotti dei *fringe benefit* per i dipendenti in una disciplina più favorevole. L'articolo 7 fa una riduzione da 10 a 5 punti per alcuni emolumenti dei lavoratori e dei dipendenti privati.

Il trattamento economico di alcune tipologie del personale della Croce Rossa è stato inserito durante l'esame in Commissione. All'articolo 10 ci si occupa dell'incremento dei fondi dello Stato per la contrattazione collettiva per il pubblico impiego e per il personale di diritto pubblico (personale prefettizio, amministrativo, civile e assunzioni).

C'è anche un'interpretazione autentica per la commercializzazione dei veicoli e poi si passa a tutte quelle norme e oneri fiscali per alcuni prodotti di tabacco, disposizioni dei valori di acquisto delle partecipazioni e all'autorizzazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti. Si estende la disciplina delle partecipate con *exemption* ai soggetti non residenti;

Le plusvalenze delle cessioni sugli immobili con interventi del superbonus e poi ci sono tutte le norme che riguardano le riduzioni o articolazioni per quanto riguarda le questioni fiscali. Sono stati introdotti poi 13,5 milioni, sempre in sede referente, per la Protezione civile e per alcuni Comuni dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo.

che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento. Questa è stata una misura introdotta proprio per salvare un comparto che in questo momento

le esigenze che provenivano soprattutto dalle persone più in difficoltà, cercando di dare risposta su tutti

che sono stati presenti in Commissione bilancio a partire dal mese di novembre (credo dal 7 novembre), quando è stata incardinata la manovra finanziaria.

Cominciamo ad avere dei segnali importanti sull'inflazione che ha caratterizzato questo periodo particolare e tutte

le misure economiche che abbiamo messo in campo anche negli anni passati, che sono stati difficili perché abbiamo vissuto il periodo oscuro della pandemia,

la guerra anche oggi alle porte dell'Europa. Non c'è un Paese europeo che oggi sta meglio di noi; siamo tutti sulla stessa barca ed è su questa barca che noi tutti dobbiamo navigare al meglio e l'Italia lo sta facendo e lo ha fatto oggi grazie innanzitutto alla stabilità politica. Desidero infatti sottolineare che la grande forza oggi di questo centrodestra e del Governo deve essere la stabilità politica, quindi la forza del nostro Paese deve essere

delle misure reali, che diano risposte ai settori maggiormente colpiti da tutta una serie di situazioni economiche congiunturali

destinando 10 miliardi di euro alla riduzione del cuneo previdenziale per i lavoratori con fasce di reddito fino a 35.000 euro,

La seconda misura è quella che riguarda la riduzione delle tasse e anche in questo caso abbiamo investito 4 miliardi di euro nella riduzione a tre aliquote

fino a 8.500 euro della *no tax area*, la detassazione dei premi di risultato, la detassazione del lavoro notturno. Per le famiglie, viene destinato un altro miliardo di euro per sostenere i genitori con figli, per favorire Abbiamo previsto l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli, il *bonus* asili nido, il fondo di garanzia sui mutui anche per le giovani coppie e soprattutto per le famiglie numerose, una misura che va

la maxideduzione per le imprese che assumono a tempo indeterminato; tra manovra finanziaria e decreto anticipi, che è un collegato, vengono destinati 150 milioni per la "nuova Sabatini" che riguarda gli investimenti strumentali; ci sono misure a sostegno delle imprese esportatrici, la proroga del fondo per promuovere la competitività,

un aspetto di responsabilità e di autenticità, anche nei confronti dei nostri giudici esterni, le Agenzie di *rating*, i Paesi europei,

Inflazione, costi energetici, incertezza internazionale sono elementi che hanno reso ancora più problematica la chiusura di una manovra di bilancio assai improba da chiudere a causa della riduzione di 33 miliardi che vanno a sottrarsi a quella parte di manovra libera che in questo caso era assai ridotta perché confacente, perché proporzionata, perché riconducibile a 20-25 miliardi. Immaginiamo cosa sarebbe stata, in termini positivi, una manovra che avesse avuto ulteriori 33 miliardi da poter spalmare su scuole,

Questa è una manovra che guarda alle famiglie, in particolar modo a quelle più numerose, e alle fasce più deboli. Con la cosiddetta Carta dedicata a te, come diceva il collega Damiani, si aiuti per l'acquisto della prima casa, aiuti per il caro energia e per il *bonus* elettricità, in particolar modo per le fasce più deboli. Cito poi la riduzione della pressione fiscale, la detassazione della produttività, detassazione dei *fringe benefit*, la detassazione del lavoro notturno, la detassazione degli straordinari nei festivi per quanto riguarda il turismo, l'esonero parziale dei contributi previdenziali per le categorie più deboli. Importanti sono i fondi messi da parte per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione con 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi nel 2025. Ma di questo parlerò di qui a pochissimo.

è l'attenzione nei confronti delle calamità naturali; lo dico da abruzzese, da persona che ha visto da vicino quanto è forte l'azione distruttiva degli eventi meteorologici degli eventi meteorologici e degli eventi sismici. Le imprese vengono incentivate, portate a stipulare

la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici sono previsti 45 milioni nel 2024 e 60 milioni nel 2025. Cito inoltre la prosecuzione dell'attività amministrativa e commissariale per gli uffici per la ricostruzione 2009 e 2016; l'attenzione particolare per la proroga dei contratti stipulati nel cratere del 2009, in deroga ai vincoli assunzionali; gli aiuti per gli eventi alluvionali; l'emergenza agricoltura. Due aspetti sono stati attenzionati con forza da questa manovra: il lavoro e la sanità, con stanziamenti ingenti, importanti e qualificanti da parte di una maggioranza che ha l'ambizione di disegnare una programmazione di legislatura, con un taglio del un taglio del cuneo fiscale di 10 miliardi e la riduzione delle aliquote Irpef da tre a due, con 4,3 miliardi. Quindi un combinato disposto di 10 miliardi più 4,3 miliardi (14,3 miliardi in tutto), che immette vero denaro nelle buste paga dei dipendenti pubblici. Mi consentirete di sottolineare l'approccio diverso e il paradigma differente che ha portato la maggioranza e questo Governo a disegnare questa manovra di bilancio, che passa da un sistema assistenziale a un sistema di premialità, anche a livello educativo, nei confronti di coloro che lavorano e non di coloro che scelgono di essere assistiti dallo Stato. Non c'è nulla di non c'è nulla di sbagliato nell'essere orgogliosamente diversi a livello politico. Questa è la strada scelta da questo Governo e questo io immagino possa essere la strada

lamentando che non ci fossero abbastanza fondi. Eppure noi abbiamo toccato i 136 miliardi di euro nel 2024 per quanto riguarda lo stanziamento sui capitoli questo credo che sia un messaggio importante. Mai uno stanziamento è stato così alto nell'ambito sanitario: 3 miliardi nel 2024, 4 miliardi nel 2025, 4,2 miliardi nel 2026, con rinnovo dei contratti, indennità per i medici per le liste attesa, potenziamento del territorio. Gli investimenti per la crescita, la ZES unica per quanto riguarda il Mezzogiorno, i contratti di sviluppo, la sicurezza nazionale. Ma questo è stato già spiegato, con precisione e con particolari ben sottolineati anche a livello numerico dai colleghi che mi hanno preceduto. Io vorrei sottolineare quanto lavoro importante sia stato fatto anche in Commissione. in Commissione. In queste lunghe giornate, che hanno visto anche delle notti di lavoro continuo, abbiamo prodotto insieme, maggioranza e minoranza, con un'azione che ha portato i relatori a svolgere un ruolo di centralità nei rapporti con i membri della Commissione, ma anche col Governo,

riassetto organico del personale appartenente alle carriere prefettizie, con la promozione dei vice prefetti a vice prefetti aggiunti;

ringrazio il nostro Presidente, il mio presidente, collega di partito, il presidente Calandrini, per il lavoro svolto in settimane di convivenza simbiotica che abbiamo avuto tutti quanti in Commissione. Ringrazio il ministro Ciriani e i suoi collaboratori, per l'azione di coordinamento con le altre forze rappresentate, sia a livello di Governo sia a livello di

pasticcini, tè e feste durate anche la notte. Io voglio dire che la nostra Commissione, maggioranza e minoranza, ha lavorato tantissimo, ha lavorato in maniera molto

del Governo, i relatori e in modo particolare i colleghi e le colleghe della Commissione bilancio e tutti noi che abbiamo cercato di portare il nostro contributo. Ci aspettavamo - lo dico subito - un po' di coraggio da parte del Governo rispetto a questo disegno di legge di bilancio e purtroppo non c'è stato. Mi dispiace dover contraddire anche le parole dei tre relatori.

Pensiamo anche alla cancellazione di 18app del Governo Renzi, solo per rimanere in tema di cultura, che ha tolto una delle poche certezze ai nostri ragazzi sul tema della formazione.

che avrebbe rimesso a sistema il Servizio sanitario pubblico, insieme al tema del PNNR, anche riguardo alle infrastrutture sanitarie. Questo, infatti, avrebbe permesso di mettere a sistema un Servizio sanitario che ha bisogno di sentire delle risposte certe e autorevoli. Lo abbiamo visto anche con lo sciopero

Dico questo con grande dispiacere, perché noi tifiamo per l'Italia, tifiamo per il nostro Paese abbiamo cercato in tutti i modi di dare disponibilità, anche in sede di Commissione bilancio, con un confronto e un dialogo, sempre pronti a collaborare e a lavorare assieme. A questo proposito voglio ringraziare la senatrice Paita, il senatore Enrico Borghi e tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo di Italia Viva anche per il lavoro che è stato fatto e i e i risultati importanti che abbiamo portato assieme alle opposizioni. Sì, perché, colleghi e colleghe di maggioranza, purtroppo i risultati più importanti li ha portati questa volta proprio l'opposizione, in un lavoro che abbiamo cercato di fare in maniera unitaria, rispondendo anche alle priorità e alle esigenze dei cittadini.

ai femminicidi. Signor Presidente, me lo faccia dire: penso anche ai due femminicidi che hanno scritto ieri un'altra pagina tragica, con la morte di una

Questi 40 milioni potevano diventare 100 se la maggioranza avesse destinato quel fondo parlamentare, che era di 60 milioni, allo stesso tema. Parlo in modo particolare anche del reddito di libertà, che abbiamo portato, grazie al lavoro congiunto di tutte le opposizioni, da 4 a 10 milioni nel prossimo triennio. cinque milioni per la realizzazione di centri antiviolenza, allo stanziamento di quattro milioni annui per finanziare i centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti. ai 20 milioni annui per la realizzazione delle case rifugio, prevedendo anche uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza disoccupate beneficiarie del reddito di libertà. Stanziamo 3 milioni annui, da qui in avanti, per iniziative formative di contrasto alla violenza domestica, anche attraverso attività di formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e di *stalking*.

e l'Alzheimer. Istituiamo sulle malattie rare un fondo per la diagnosi avanzata, stanziando un milione di euro e stanziamo un ulteriore milione per i test di profilazione genomica dei tumori. Insomma, è un risultato importante che, per le poche risorse e per il poco dialogo che siamo riusciti a instaurare con la maggioranza e con il Governo, abbiamo portato a casa come opposizioni. Rifinanziamo il fondo per l'Alzheimer e le demenze, che si sarebbe esaurito quest'anno, se non ci fosse stata l'approvazione di questo emendamento. Lo rifinanziamo con 5 milioni di euro per il 2024 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, proprio per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da questa malattia. Insomma, Presidente, sono tutti temi che dovrebbero essere prioritari nell'agenda del Governo per i prossimi anni. Questo è avere lungimiranza, questo è pensare al bene del Paese e soprattutto pensare che, con le poche risorse che abbiamo, dobbiamo individuare un'agenda politica fatta di priorità. Signor Presidente, vorrei terminare, nei pochi minuti che mi rimangono a disposizione (perché cercherò di stare dentro i dieci minuti), minuti), soffermandomi ancora di più sul tema del contrasto alla violenza di genere. Poi altri temi saranno affrontati nella discussione generale sulla legge di bilancio dagli altri miei colleghi e colleghe del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. Sul contrasto alla violenza di genere quest'Assemblea poche settimane fa ha votato, fortunatamente all'unanimità, l'inasprimento delle pene e il rafforzamento del codice rosso. Ma noi, colleghi, ne usciamo fuori non solo mettendo fondi strutturali su questo tema, ma soprattutto facendo un investimento su politiche di prevenzione

ha ripercussioni positive o negative sulla vita quotidiana dei cittadini. Quando parliamo di questi temi, guardiamo a tutto il Paese. Se vogliamo cambiare l'agenda politica, ma soprattutto se vogliamo segnare un salto culturale della nostra società, dobbiamo cominciare a parlare di questi questi temi. E parlare anche in quest'Aula - e chiudo con questo - di amore, di felicità e di gentilezza significa saperci rispettare di più tra di noi, perché noi siamo avversari politici, ma non siamo nemici, e dobbiamo parlare

il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso: amarsi. Affrettiamoci ad amare e soprattutto ricerchiamo la felicità ogni giorno. Spero che anche questo tema possa combattere realmente una società sbagliata e violenta, che non contrasta la violenza di genere ogni giorno. *(Applausi)*.

quella di bilancio è la legge più importante dello Stato, con la quale non solo un Governo decide di allocare le risorse per le necessità del Paese, del Paese, ma si stabilisce la visione che il Governo e il Parlamento vogliono dare alla società. Per questo si chiama manovra, perché deve indicare la rotta, la direzione di marcia, una destinazione comune.

prevede infatti di indebitare i cittadini italiani facendo un taglio delle tasse solo provvisorio, non investe sull'economia, sull'istruzione e soprattutto sulla sanità, che è la vera emergenza nazionale del Paese, come dimostrano le liste d'attesa del nostro servizio sanitario nazionale.

indicando alcune priorità chiare, tra cui appunto la sanità. Avevamo proposto un aumento delle risorse della sanità pubblica, l'aumento del 30 per cento dei salari degli infermieri e dei medici, l'eliminazione del taglio delle pensioni, un piano di assunzione di medici e di infermieri e l'attivazione di un piano di 2 miliardi di euro per ridurre le liste d'attesa. Non me ne vorrà il senatore Liris, al quale mi lega una stima personale anche per l'attività professionale che svolge, ma citare i 136 miliardi di euro del 2024 come la più alta cifra mai spesa dallo Stato italiano significa dire il vero, ma non ha senso, se è avulso dal contesto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione. Infatti, con 136 miliardi di euro nel 2024 si compra ciò che si comprava con 116 miliardi di euro nel 2019. Allora, se vogliamo dire che l'Italia investe nella sanità, lo dobbiamo dire al netto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione, altrimenti non ha senso. Le nostre proposte avevano un costo complessivo di 10 miliardi di euro e, come veniva citato precedentemente, sarebbe bastato adottare il MES sanitario MES sanitario (non il MES nazionale, sul quale so che c'è un po' di confusione) per trovare le risorse per poterlo fare. Sull'istruzione, avevamo proposto la sperimentazione contro la dispersione scolastica nelle aree di crisi sociale e il potenziamento delle borse di studio per studenti universitari per un costo complessivo di due miliardi. Sul avevamo chiesto la conferma del taglio del cuneo fiscale già previsto e le aliquote agevolate per i prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile, per un costo complessivo di 10 miliardi. Sulle avevamo chiesto l'attuazione del *family act* per il sostegno alle famiglie e al lavoro femminile e una fiscalità di vantaggio per il rimborso delle spese per i figli, per un costo complessivo di due miliardi. Sull'industria

misure precise, realizzabili, per un costo complessivo di 24,4 miliardi di euro. Tutto questo non è stato accolto, senza nemmeno una discussione politica. E qui arriviamo a un errore di metodo, che per noi è grave e di cultura politica: continuare a svilire le prerogative di tutto il Parlamento. Questo Governo dimostra, ancora una volta, di avere paura del Parlamento, ma ciò che colpisce di più è che abbia paura della sua maggioranza. È un vero peccato, perché molti emendamenti (noi di Azione ne avevamo proposti 92, ma tutti gli emendamenti delle opposizioni erano 2.700) miravano a migliorare la manovra e avrebbero potuto essere recepiti dai relatori della maggioranza. Permettetemi di ringraziare i senatori Testor, Liris e Damiani, il Presidente della Commissione bilancio Calandrini e tutto il personale della 5a Commissione per il lavoro svolto. Tutti i componenti hanno cercato di fare del loro meglio, ma che senso ha discutere fino a tarda notte in Commissione, se il Governo toglie la possibilità di svolgere la mediazione, il dialogo e l'ascolto, che sono l'essenza dell'arte della politica e della dialettica parlamentare? Che senso ha discutere di tutti gli emendamenti, alcuni dei quali avrebbero potuto essere accolti anche dai relatori di maggioranza, se non c'è la disponibilità da parte del Governo? E questa disponibilità non c'è perché la paura non è tanto del Parlamento in quanto tale, ma è della maggioranza parlamentare e questo svilisce le prerogative di tutti. È un vero peccato, perché penso agli emendamenti che avremmo potuto portare a casa tutti insieme come vittorie comuni. Penso agli emendamenti sulla disabilità per le indennità per i sordociechi. Penso agli emendamenti per favorire l'acquisto di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone disabili. Penso agli emendamenti sui fondi per i piccoli Comuni delle aree interne o dei Comuni montani sotto i 3.000 abitanti, che devono trasferire le quote dell'IMU sulle seconde case al Fondo di solidarietà nazionale e non possono utilizzarle come risorse proprie per finanziare i servizi. Penso all'emendamento sulle gare Consip per la sanità digitale, al rimborso delle spese per favorire il voto dei fuori sede (poi non lamentiamoci del fatto che ogni volta l'indice della partecipazione al voto scende). Penso all'inquadramento di 4.000 volontari del servizio civile universale per la ricostruzione post-alluvione dell'Emilia-Romagna. Una nota positiva - lo voglio che tutte le opposizioni hanno avuto nell'idea di usare le risorse del fondo parlamentare (40 milioni di euro, di cui 20 di spesa corrente e 20 in conto capitale) non per mancette elettorali, ma per scegliere di dare una priorità che voleva essere anche un messaggio chiaro al Paese: destinare tutte queste risorse contro la violenza di genere, per il finanziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e del reddito di libertà, offrendo al Paese un gesto di serietà, responsabilità e unità. Sono convinto che questo sia un successo non solo delle opposizioni, ma di tutto il Parlamento, perché so che questi emendamenti sono condivisi anche dalla maggioranza. In conclusione, signor Presidente, per restare nei termini, la nostra contrarietà è nel metodo e nel merito. Rischiamo di approvare una legge di bilancio senza visione, senza rotta, senza manovra e, ciò che è più preoccupante, con un metodo che purtroppo continua a svilire le prerogative di tutto il Parlamento.

Signor Presidente, senatori, in quest'Aula discutiamo di una legge di bilancio che si presenta come un punto di equilibrio nel delicato compito di sostenere la crescita economica, le famiglie e il settore pubblico, pur mantenendo la sostenibilità finanziaria. In questi tempi turbolenti, ci troviamo a bilanciare la prudenza finanziaria con l'audace necessità di promuovere la crescita e il benessere del nostro Paese. Al di là di quelle che possono essere le narrazioni di parte, la legge testimonia un percorso difficile, gravato da situazioni precedenti complesse - lo diceva prima il collega Damiani, che ringrazio insieme agli altri relatori, alla Commissione e al presidente Calandrini e da precedenti decisioni che seguivano proprio quelle situazioni difficili, in particolare, i crediti d'imposta dei *bonus* edilizi e i maggiori interessi passivi sul debito pubblico.

prorogarlo di qualche mese per chiudere i lavori che sono già in corso per evitare problemi ai condomini e alle imprese - ma comunque continuano i *bonus* edilizi come il sismabonus, l'ecobonus, i *bonus* sugli elettrodomestici e gli altri *bonus* dal 70 al 50 per cento.

e sostenga le famiglie e il settore pubblico. Questa legge, con saggezza e precisione, dirotta le risorse dalla spesa improduttiva a quella sociale; riduce le tasse, com'è nel DNA e nella politica di Forza Italia, stimolando la crescita e sostenendo le famiglie italiane. Viene dimostrato un impegno concreto nei confronti dei nostri lavoratori della sanità e dell'intera pubblica amministrazione. Si equilibra il sistema pensionistico con la protezione dei diritti dei lavoratori e si sostengono le madri lavoratrici. Le misure di sostegno introdotte proprio per le madri lavoratrici sono un passo significativo nell'affrontare un problema enorme, la sfida demografica del nostro Paese, e nell'offrire anche un aiuto concreto alle donne e alle famiglie. Si prendono provvedimenti significativi per il rilancio del Mezzogiorno, dalla riduzione del cuneo previdenziale alla revisione dell'Irpef. Ogni misura è stata ponderata per massimizzare il beneficio per i lavoratori del Sud. La manovra dimostra quindi un impegno concreto e la volontà di rinnovare i contratti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al personale medico sanitario. La destinazione di risorse aggiuntive per il finanziamento della spesa sanitaria è un passo fondamentale per garantire servizi pubblici efficienti, in particolare proprio nelle Regioni del Sud, dove questa necessità si fa più pressante. Permettetemi ancora di più di focalizzare la mia attenzione sugli effetti positivi che questa manovra avrà per il Sud del nostro Paese. Il Mezzogiorno nel suo complesso si erge come il principale beneficiario di tale manovra. I 10 miliardi di euro destinati al cuneo previdenziale per i redditi fino a 25.000 euro, con la riduzione di sette punti percentuali e di sei punti per i redditi fra 25.000 e 35.000 euro rappresentano un miglioramento significativo per molti redditi dei lavoratori del Sud. Anche la revisione delle aliquote Irpef avrà un impatto notevole sui redditi bassi, quindi ne beneficerà direttamente il Mezzogiorno. La legge di bilancio stanzia fondi significativi, com'è stato detto per il credito d'imposta sui beni strumentali, per la ZES unica del Mezzogiorno, e questa è stata una svolta per il rilancio economico del Sud, un'idea del ministro Fitto. La ZES unica è destinata a far crescere la produzione delle imprese meridionali, contribuendo all'aumento dell'occupazione, come i fondi stanziati con la Sabatini, che daranno alle imprese la possibilità di dotarsi di nuove attrezzature, di nuove tecnologie anche per implementare i nuovi processi produttivi. Non dimentichiamoci gli investimenti infrastrutturali, in particolare i 780 milioni di euro destinati al ponte sullo Stretto, un'opera che promette di generare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. È giusto quindi che ci sia anche un contributo da parte delle Regioni direttamente interessate. Inoltre, accolgo con favore il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e le norme che incidono direttamente sui territori. Sono orgoglioso del finanziamento all'università della Calabria, tre milioni e mezzo di euro in tre anni, per lo sviluppo di personale esperto in medicina digitale, per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia in grado di elevare il livello della prestazione sanitaria del Servizio sanitario regionale, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi. Cito poi il finanziamento al Comune di Caivano, cui è destinato un importo fino a 15 milioni di euro in favore di una nuova area di crisi industriale. ricordo l'integrazione dell'Agenda Sud e il rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni meridionali attraverso assunzioni in deroga, che sono passi fondamentali per promuovere lo sviluppo e l'efficienza ammnistrativa del Sud Italia. Sempre in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, viene estesa a tutte le amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Calabria la disposizione che autorizza le amministrazioni interessate da fenomeni migratori, anche in deroga, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientrati nei percorsi di inclusione. Si prevede poi la proroga al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione della Regione siciliana che consente la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo. Sono misure che dimostrano l'attenzione continua di questo Governo verso le problematiche del Mezzogiorno. quindi di dire che questa legge di bilancio non è solo un documento finanziario, ma è un documento di intenti, un manifesto di speranza e progresso per il nostro Paese, una dichiarazione delle nostre priorità e dei nostri valori, per quanto riguarda la maggioranza e Forza Italia, che pone al centro del benessere dei cittadini la prosperità del Mezzogiorno. Con questa legge proclamiamo oggi il nostro impegno per una Nazione più giusta, più forte e più unita.

la legge di bilancio 2024 è l'ennesimo provvedimento vuoto di contenuti e soprattutto di soluzioni. Negli interventi che mi hanno preceduto abbiamo risentito la solita cantilena e il solito piagnisteo di risorse scarse,

che le misure che oggi il Governo ci propone e che il Parlamento dovrà approvare avranno sulla vita delle imprese e dei cittadini. Gli impatti sono devastanti. sono devastanti. I bollettini economici che stiamo leggendo in queste settimane (di Istat, OCSE, Banca d'Italia) fotografano una realtà diversa da quella che sentiamo ogni giorno in TV e leggiamo sui giornali *(Applausi)*, e sentiamo la cantilena anche qui in Parlamento.

Le crisi dell'ultimo decennio non vi hanno insegnato nulla perché, oggi come allora, la spesa la considerate solo un costo da contenere e tagliare a prescindere, senza considerare il suo possibile ruolo di motore della crescita. Keynes per voi continua ad essere un perfetto sconosciuto.

misura anche voi l'avete utilizzata, prorogata più volte, e adesso la utilizzate per nascondere solo le vostre incapacità. Il debito pubblico per voi è solo una passività da ridurre non con la crescita economica, ma con i tagli e le privatizzazioni, ignorando gli effetti che poi producono quei tagli e quelle privatizzazioni. Il ritorno del *surplus* primario il ritorno della flessibilità e della precarizzazione del lavoro sono peraltro l'esatta conferma del peggior neoliberismo austeritario. I risultati sono evidenti, come dicevo: una produttività stagnante, una crescita dello zero virgola, tagli alla spesa pubblica e riduzione degli investimenti e della spesa sociale. Il mancato sostegno alla domanda, la rinuncia a sostenere i salari divorati dall'inflazione e la decisione di non contrastare la povertà e non salvare il Servizio sanitario nazionale stanno ulteriormente indebolendo l'economia, lo Stato sociale e la sostenibilità del Paese. State anche sottovalutando le implicazioni del calo della domanda, ma soprattutto dei consumi, delle famiglie. Aggiungo anche che la mancata possibilità di accesso al mercato del credito, sia per le imprese sia per le famiglie, può avere effetti devastanti in un Paese come il nostro, ad alto debito. Avete programmato un avanzo primario strutturale del 3,2 per cento, che equivale a circa 50 miliardi di tagli che dovete fare nei prossimi anni. Altro che retorici richiami alla crescita, quando questa è pari allo zero, o proclami per rafforzare il sistema sanitario e sostenere la transizione ecologica. Dimenticate che le regole di bilancio sono un mezzo per raggiungere un fine e non un fine in sé. Se il fine è promuovere la crescita,

della politica economica del nulla che state portando avanti, con la quale avete rinunciato a tracciare un percorso verso l'innovazione, verso la riconversione di quell'impianto e soprattutto verso la diversificazione industriale di quel territorio, oltre che di quella economica, sociale e culturale. Per mantenere il debito pubblico su un sentiero sostenibile, quindi, è necessario tracciare nuove rotte, razionalizzando eventualmente la spesa o sostenendo nuove spese produttive, ad alto valore aggiunto. L'assenza di una politica economica e la crescita utopistica dell'1,2 per cento del PIL che avete programmato, quando oggi sappiamo benissimo che sarà al massimo dello 0,7 per cento è l'esatto contrario di quello che state dicendo sulla crescita economica del Paese. Questo differenziale produrrà un vuoto di bilancio, che vi costringerà, a partire da giugno, ad approvare una manovra correttiva. Ve lo stiamo già dicendo. Avete portato avanti per mesi la politica del piagnisteo per le risorse che non c'erano. Noi abbiamo avuto il coraggio di presentarvi una contromanovra, in cui vi abbiamo detto dove andare a prendere circa 35 miliardi. Vi sintetizzo alcune di queste misure: la tassazione sugli extraprofitti bancari, annunciata in pompa magna, in conferenza stampa, e poi ritrattata; il recupero, in questo caso del vero buco di bilancio, generato da quella falsa tassazione sugli extraprofitti energetici che ha lasciato che ha lasciato Draghi e che voi non avete recuperato; la rinuncia ad estendere il contributo di solidarietà anche ai settori farmaceutici, assicurativo e bellico. Non avete razionalizzato i sussidi ambientalmente dannosi, ci sono oltre 22 miliardi su cui si poteva agire. Non avete aumentato la tassazione sulle transazioni finanziarie, oltre poi a non aver aumentato quella sull'economia digitale. Per non parlare poi della lotta all'evasione fiscale, cui avete completamente rinunciato, introducendo uno strumento, il concordato preventivo biennale, che sarà un fallimento, per come voi stessi lo avete certificato, avendo stimato di poter riscuotere oltre 200 milioni di euro. Presidente, è sempre più commovente la superficialità del Governo.

vestendo gli improbabili panni dell'economista, quando ha fatto riferimento al rimbalzo del gatto morto.

peccato che la crescita economica che abbiamo realizzato ci abbia permesso di essere la locomotiva d'Europa.

Adesso invece, secondo gli ultimi dati economici che non sto qui a sintetizzare, il gatto (nero) voi lo avete stecchito su un binario morto. Signor Presidente, concludo

«Vana è la gloria di chi cerca la fama solo nel luccicare delle parole». *(Applausi)*. Grazie Presidente. disegno di legge di bilancio che stiamo per votare si conferma ancora una volta la grande unità di intenti e di azione che caratterizza la nostra maggioranza. maggioranza. Ci rendiamo conto che questo causa non poche preoccupazioni e malumori, espressi in polemiche sterili e maldestri tentativi di generare disaccordi da parte delle opposizioni. La nostra unità rappresenta però uno dei principali punti di forza di questo Governo, che prosegue, anche con il fondamentale strumento di programmazione economica al nostro esame, sulla strada segnata fin dall'inizio della nostra legislatura, ovvero il sostegno alle famiglie, ai redditi medio-bassi e alle imprese, ancora una volta dimostrando come ciò che conta per noi siano solo le esigenze del Paese reale, senza menzionare gli ingenti investimenti in termini di infrastrutture, nonostante il momento e la prudenza della manovra, perché una finanziaria senza investimenti non ha visione. Uno dei fronti principali su cui agiamo è il lavoro, attraverso un pacchetto di misure che prevede interventi variegati, utili a offrire nuove opportunità e liberare nuove risorse in un mercato che che finora è stato soffocato da tassazione, da burocrazia e da decisioni politiche miopi e vessatorie nei confronti degli operatori, siano essi datori di lavoro o lavoratori, che finora hanno avuto solo l'effetto di contrarre l'occupazione e accrescere la povertà. Certo, anziché limitarci a distribuire sussidi improduttivi, che sarebbe stato molto più facile anche per noi, stiamo costruendo le basi migliori per creare sviluppo e posti di lavoro, che è quello che abbiamo promesso fin dal nostro insediamento e su cui stiamo puntando già da tempo. Ecco allora che alle misure varate già nei mesi scorsi questa manovra ne aggiunge altre altrettanto importanti. Parto dal *bonus* assunzioni, un provvedimento voluto in particolare dalla Lega, per il quale le agevolazioni per le assunzioni non consistono più in una semplice decontribuzione INPS, com'è stato finora, ma in una maxideduzione del costo del lavoro cento, che aumenta e può arrivare fino al 130 per cento per i nuovi assunti, nel caso di categorie svantaggiate, come gli *under* 30, i percettori di reddito di cittadinanza o le persone con disabilità. strumento riuscirà a moltiplicare gli occupati, offrendo nuove opportunità alle imprese di creare lavoro e ai lavoratori di trovare un impiego. Sempre nell'ottica di aiutare il lavoro, manteniamo il taglio del cuneo fiscale del 7 e del 6 per cento, rispettivamente per i dipendenti fino a 25.000 e destinando a questa misura 10 miliardi, con aumenti in buste paga che vanno dagli 80 ai 100 euro al mese, che per i nostri avversari, evidentemente abituati a introiti ben più ghiotti, sono briciole, ma che invece per milioni di lavoratori che ne continueranno a beneficiare rappresentano un aiuto importante per poter arrivare a fine mese con un po' più di serenità. Continuiamo poi a detassare i premi aziendali e i *fringe benefit* fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico, alzando da 258 a 1.000 euro la soglia esentasse per tutti gli altri; beneficio che, se usato in maniera intelligente da aziende e lavoratori, investendo sul *welfare* aziendale, può dare un ulteriore respiro sia al tessuto imprenditoriale sia alle famiglie dei lavoratori. Rendiamo poi strutturale un'altra misura particolarmente utile al popolo delle partite IVA, il cosiddetto bonus 800, cioè l'indennità di continuità reddituale per gli autonomi, che, come sappiamo, agisce da ammortizzatore sociale per chi registra un forte calo di fatturato, entro

Come intervento di grandissimo impatto, dopo anni di immobilismo, mettiamo finalmente mano ai contratti del pubblico impiego, con un rinnovo da 5 miliardi per la pubblica amministrazione e di 2,5 miliardi per il personale medico sanitario, fondi che in buona parte confluiranno in aumenti retributivi. Credo che questo possa essere un grande successo

tante misure di valenza sociale: manteniamo la *social card*; prevediamo il *bonus* per le mamme lavoratrici con almeno due figli, che vedranno aumentare la busta paga al netto; diamo un respiro alle donne sulla conciliazione vita-lavoro, con il congedo parentale e il *bonus* per gli asili nido; istituiamo il fondo per il contrasto al disagio abitativo e aumentiamo di 282 milioni di euro il fondo per la prima casa. casa. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti che inciderà positivamente sulla vita delle famiglie. Voglio chiudere con le misure previste per il Sud, in particolare il *bonus* macchinari per l'acquisto di beni strumentali per gli stabilimenti produttivi collocati nel Mezzogiorno, misura che si aggiunge all'importantissimo quadro di provvedimenti introdotto dal decreto Sud.

credo che il Governo raggiungerà ottimi risultati, nonostante il momento e la prudenza del caso. Voglio quindi ringraziare il presidente Meloni, i vice presidenti Salvini e Tajani, il ministro Giorgetti,

Presidente, noi pensiamo che la manovra di bilancio che il Governo Meloni ha imposto faccia male al nostro Paese: è una manovra cinica, senz'anima, fatta di tagli, di inganni e di mance, di giochi di prestigio e di sotterfugi a danno di tutti, ma soprattutto di chi è più debole, di chi è senza difesa. Non c'è protezione in questa manovra per chi è in difficoltà. Questa, Presidente, è la legge di una destra che non ha nulla di sociale, ma è una destra delle diseguaglianze e il cui sottotesto è il seguente: ognuno si arrangi da solo

Avete imposto un disegno di legge di bilancio senza discussione, mortificando il Parlamento, annunciando tempi *record*, invece poi arrivando sull'orlo dell'esercizio provvisorio, che è come dire sull'orlo del dissesto. Ci avete condotto a questo perché siete divisi, anche se non lo date a vedere, perché siete arroganti - e questo si comincia a vedere e perché siete sotto scacco dei mercati e delle agenzie di *rating*, e questo si vede benissimo. *(Applausi)*. La vostra ossessione è stata non sfigurare davanti alla finanza internazionale: avete fatto una manovra che forse potrà piacere a qualche circuito d'*élite,* ma che sicuramente non potrà piacere agli italiani. In questa manovra non ci sono investimenti; è una manovra cieca, senza un'idea di futuro. Non c'è niente per il lavoro, quello da difendere e quello da creare; non c'è niente per le imprese, che sono la nostra spina dorsale, altro che la vostra retorica sul *made in Italy*. Non c'è nulla per la crescita, mentre il Paese è fermo, è in stagnazione. È una visione d'Italia distorta, che ingigantisce disparità e discriminazioni. Con questa manovra voi mettete a rischio il Servizio sanitario pubblico nazionale. Continuate a riempirvi la bocca dicendo di aver aumentato i fondi, ma è solo propaganda e lo sapete bene, perché i vostri stanziamenti per la sanità non riescono a compensare né l'aumento dell'inflazione, né il crollo del prodotto interno lordo e questo significa che la sanità pubblica sarà tagliata. Voi lo sapete, ma non siete intervenuti. Continuate a raccontare la favola del *record* di risorse e invece lasciate che venga colpita, che venga smantellata la sanità pubblica. Eppure, come sapete, nel nostro Paese ci sono migliaia e migliaia di persone che non riescono a curarsi, che non possono curarsi perché i tempi di attesa sono troppo lunghi, anche per le visite urgenti, anche per gli esami oncologici, quelli che sono indispensabili, quelli che significano la vita. Tante persone rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi necessari per andare dal privato, per saltare la fila. fila. Presidente, noi rifiutiamo questa idea di società dove chi ha i soldi può curarsi e dove chi invece non li ha è lasciato solo

e dei lavoratori dentro la grande trasformazione digitale, ecologica, tecnologica che viviamo e che rischia di scaricarsi sui più deboli. In Italia ci sono milioni di lavoratrici e di lavoratori poveri che si spaccano la schiena e l'anima, che fanno più occupazioni contemporaneamente per arrivare alla fine del mese, per provare a mettere qualcosa da parte, ma in questa legge nulla. Non c'è nulla perché questa destra ha voluto affossare la nostra battaglia di civiltà per il salario minimo, tradendo l'attesa di oltre 3,5 milioni di lavoratori poveri. Perché sotto i 9 euro l'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. *(Applausi)*. Oggi c'è in Italia una miriade di persone costretta a lavorare per 4 o 5 euro l'ora, che non riesce, non può riuscire a pagare bollette, affitti, un mutuo. In questa legge non c'è niente contro il carovita. Ci sono però

penali miliardarie come ai tempi del Governo Berlusconi. Mi riferisco - tutti lo sapete - al Ponte sullo Stretto, un'opera sbagliata che impatta su un ecosistema fragilissimo e che nessuno effettivamente vuole, all'infuori del capriccio del vice *premier* Salvini, tanto che ci sono manifestazioni anche con la presenza di sindaci siciliani che chiedono di fermarsi. E invece no, la propaganda del Governo non si ferma. E dove prende il Governo i soldi per far partire gli appalti del Ponte, per alzare gli stipendi ai *manager* del Ponte, come avete già fatto? Prende i soldi da chi è più debole: voi togliete miliardi di risorse già stanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sono risorse per la lotta alla povertà, per l'inclusione sociale, per la casa, per l'acqua, per l'edilizia popolare, per le infrastrutture territoriali, per i lavori pubblici, per il lavoro. Ebbene, da oggi quelle risorse non ci sono più e questo è pazzesco. Presidente, non c'è nulla in questa legge sulle calamità naturali. Non c'è praticamente nulla sui crateri sismici. Voi voltate le spalle a intere comunità di un entroterra senza servizi a cui avete negato la zona economica speciale (ZES), a cui state negando la possibilità di una ripartenza. Non c'è futuro in questa manovra, non c'è nulla per le nuove generazioni, nulla per la scuola, per l'infanzia, nulla per gli asili nido. Tranne in realtà per un unico asilo nido, uno soltanto, quello del Comune di Montereale Valcellina, vicino

Non c'è nulla contro la povertà educativa, nulla per l'indennità di discontinuità ai lavoratori della cultura, tra i più precari, che noi avevamo pensato come strumento di *welfare* universale e voi avete mortificato a mancia offensiva per pochi, a fronte di molti tagliati fuori. nulla per l'università, la ricerca e il diritto allo studio; nulla per dare attuazione al contratto di ricerca, che è stata una conquista storica contro il precariato. nulla per il reclutamento di nuovi ricercatori, nulla per permettere alle ragazze e ai ragazzi delle famiglie che non sono agiate di continuare a studiare, di scommettere sul proprio talento, di inseguire i propri sogni. Di quale merito parlate allora? Voi che avete inserito la parola «merito» nel titolo di un Ministero poi permettete solo ai ricchi di studiare. La vostra è una gara truccata. Non avete rifinanziato il Fondo per gli affitti, eppure sapete che ci sono studenti in tenda da mesi negli atenei di tutta Italia che protestano, perché è diventato impossibile riuscire a pagare le spese di un posto letto, quelle della mensa, dei libri, dei trasporti, in un Paese come il nostro dove le tasse universitarie sono tra le più alte d'Europa e dove non esiste un *welfare* studentesco. Il nostro è un Paese dove i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi - lo dice la nostra Costituzione - devono poter andare avanti e invece si vedono preclusa la possibilità di una borsa di studio per mancanza di risorse, dove la dispersione e l'abbandono scolastico e universitario sono un macigno troppo grande per la vita di troppi ragazzi. Non c'è niente in questa legge che parli di emancipazione e niente che parli ai bisogni e alle aspettative che sono fuori da quest'Aula; fuori di qui c'è un mondo che avete tradito. Avevate promesso in campagna elettorale più pensioni e invece attaccate le pensioni, in particolare quelle delle donne e dei dipendenti pubblici. Non c'è nulla per la non autosufficienza e questo è tremendo. Alzate l'IVA sui beni di prima necessità come gli assorbenti o i pannolini per i neonati, mentre l'avevate abbassata sulla chirurgia estetica. Il vostro è un mondo fuori dalla realtà Presidente, ho concluso - è propaganda fasulla, carta straccia. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti senza nemmeno discuterli, ma noi continueremo a batterci per un'idea di Paese alternativa alla vostra, dove nessuno sia lasciato solo, dove tutti abbiano la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita.

tutti i rappresentanti dei partiti che ne fanno parte, sia di opposizione che di maggioranza, e in particolar modo i tre relatori.

Purtroppo però vorrei segnalare un fatto increscioso che prima il senatore Liris ha tentato di accennare. di accennare. Alcuni quotidiani hanno voluto fare un attacco diretto al Vice Presidente della Commissione, pensando di essere spiritosi, ma hanno

Questo - secondo me - è un fatto molto grave che non deve più verificarsi. Qualcuno, dai banchi dell'opposizione, diceva che il Governo lavorava col favore delle tenebre per scrivere questa manovra. Però io, sommessamente, vorrei ricordare che negli anni in cui noi eravamo all'opposizione e qualcun altro - penso al Partito Democratico, ma soprattutto ai 5 Stelle - era al Governo, le leggi di bilancio non è che eccellessero per organizzazione e tempistiche. Se dobbiamo guardare alla legge di bilancio del 2021, il provvedimento è arrivato al Senato il 29 dicembre, praticamente a un giorno dalla scadenza e proprio a un passo dall'esercizio provvisorio che da sempre, da quando stiamo trattando il tema della manovra, il senatore Patuanelli minaccia come uno spauracchio continuo e permanente. Sempre nella discussione della il Presidente della Commissione pentastellato si diceva mortificato per il fatto che la Commissione non fosse riuscita a dare il mandato al relatore,

Potrei continuare con tanti altri esempi. Quindi, io non vorrei parlare di questo, cioè avere un confronto tra maggioranza e opposizione su questi temi, perché secondo me non ne uscite bene. bene. Se vogliamo fare un discorso serio e costruttivo sulle fragilità dei Regolamenti parlamentari, sulle carenze nell'ammodernare la macchina dello Stato portandola verso l'efficienza e la semplificazione, superando il superando il monocameralismo alternato, noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a discutere di questi temi, perché abbiamo il senso dello Stato. Il Governo sta mettendo in campo degli interventi costituzionali per migliorare la macchina organizzativa. Cambiare il bicameralismo paritario, rafforzare la stabilità del Governo e il sistema delle garanzie possono aiutare l'Italia ad essere più libera, più forte e più prospera, ed è in questa direzione che il presidente Giorgia Meloni sta guidando il Governo dell'Italia. Il provvedimento di cui stiamo disquisendo e che ci accingeremo a votare in questi giorni ha subito ha subito pochissime variazioni rispetto all'approvazione fatta il 16 ottobre nel Consiglio dei ministri. I principali I principali temi e punti di riferimento con cui è stata scritta la manovra sono la prudenza, la responsabilità e soprattutto il senso di realtà con cui stiamo vivendo. C'è stata una completa discontinuità rispetto al passato. È una questione di mentalità, di approccio diverso che abbiamo noi nell'affrontare i temi che riguardano i cittadini italiani.

l'Italia sta andando bene, perché la Borsa affari sta ottenendo risultati che non faceva da anni il PIL italiano cresce di più di quello tedesco e francese *(Applausi)*, che devono essere i nostri punti di riferimento, il *benchmark*. Nella legge di bilancio, come promesso agli italiani - per noi per le promesse vanno mantenute abbiamo ridotto il cuneo fiscale, perché riteniamo che il fisco debba essere equo. Quindi sono stati messi 10 miliardi in manovra Il tutto sempre in un contesto difficile. È inutile che ci dite che noi ci aggrappiamo alle solite congiunture internazionali, perché queste congiunture ci sono e con esse dobbiamo fare i conti.

È un'eredità pesantissima quella che i Governi giallorossi ci hanno lasciato. Fa specie poi leggere che l'INPS di recente ha chiarito che il provvedimento del superbonus ha attivato solo 1.500 contratti di lavoro. Se facessimo una semplice e banale

presente. Non citerei tanto Keynes, ma chiederei alla Guardia di finanza quanti sono i miliardi

Poi, sempre dei banchi dell'opposizione, signor Presidente, ci viene detto che noi non abbiamo una visione, che questa manovra non sostiene l'economia. Bisogna avere una visione complessiva. Non possiamo analizzare solo la manovra del 2024, perché la manovra poi ha dei collegati. Ad esempio, abbiamo appena votato il decreto fiscale. Poi, grazie anche al Governo Meloni, cara opposizione, siamo riusciti ad andare a

potranno utilizzare, per il rilancio dell'economia, più di dodici miliardi. Signor Presidente, la manovra non va dunque vista solamente coi conti legati alla legge di bilancio 2024, ma va analizzata nel suo complesso, perché un Governo, uno Stato che è stratega, deve saper muovere su più livelli. I relatori hanno raccontato ed elencato tutti gli obiettivi che questa manovra ha raggiunto, ma ci tengo a raccontare un obiettivo che ho seguito io personalmente, insieme ai colleghi Nocco, Tosato e Pirovano. l'obiettivo di non far passare un terribile Natale a centinaia di famiglie che lavorano nei poligrafici. Siamo riusciti a trovare le risorse, risorse per portare al pensionamento diverse centinaia di lavoratori nel settore dei poligrafici. Questo obiettivo lo abbiamo raggiunto con un lavoro di squadra nel centrodestra, con l'aiuto anche dell'UGL, che ci ha supportati, ma mancando qualche attore importante nel settore sindacale. La CGIL, ad esempio, per questo settore non si è stracciata le vesti, non ha fatto attività di *moral suasion*. Forse era più intenta a firmare contratti di lavoro che sono ben al di sotto i 9 euro, piuttosto che sostenere lavoratori in difficoltà e che rischiavano di passare un Natale terribile. Presidente, prima il collega Lombardo ha parlato del fatto che noi ci vantiamo di aver raggiunto il *record* storico in valore assoluto e, giustamente, ci ha fatto notare che esiste l'inflazione. Intanto, c'è da dire che l'inflazione, col Governo Meloni, si è ridotta e di gran lunga. Ciò vuol dire che l'attività fatta paga e che i cittadini italiani possono stare più sereni. Ma non possiamo analizzare quanto detto dal collega Lombardo, signor Presidente, in modo così

di legge di bilancio getta le basi per rilanciare la nostra Nazione. Noi di Fratelli d'Italia siamo molto ottimisti che questa sarà una legge di bilancio, che

sul valore e il senso che ha questa discussione, che dovrebbe essere una delle discussioni più alte del Parlamento, perché stiamo discutendo della legge di bilancio e quindi delle scelte che si fanno per il Paese. Sono abituata, per la mia storia personale, a ragionare sempre su che cosa si prospetta per il Paese, a partire da un tema che si chiama il lavoro: se dalle scelte che si fanno i lavoratori e le lavoratrici, ma da questo punto di vista anche la qualità delle imprese, avranno degli effetti positivi oppure no. Vorrei partire da un tema su cui, come Assemblea, non molto tempo fa ci siamo tutti insieme impegnati. Discutevamo dell'ennesima strage sul lavoro abbiamo detto che quella era una priorità per il nostro Paese e per il Parlamento, perché quasi tre morti al giorno sul lavoro non sono sopportabili. Vorrei dire a tutti noi che gli infortuni quest'anno hanno già raggiunto il mezzo milione. Allora forse uno si aspetta che nella legge di bilancio ci siano delle risposte non emergenziali, perché la legge di bilancio non è l'ennesima emergenza su cui decretate ogni giorno, ma di prospettiva. Mi Mi sovviene che c'era un emendamento che proponeva, sulla base delle risorse già esistenti all'INAIL - e quindi senza neanche pretendere che ci fossero chissà quali investimenti di provare a costruire una relazione con quelle imprese che, occupandosi di digitale, di strategie della robotica e di nuova transizione digitale, investissero sul fatto che il digitale fosse utilizzato per garantire la sicurezza dei lavoratori. Una piccola cosa di prospettiva, che però aveva al centro il fatto che per noi, per il Parlamento italiano, difendere la vita dei lavoratori dovrebbe essere un obiettivo quotidiano. Eppure, avete detto di no. Guardate: ho anche il sospetto che non l'abbiate neanche letto l'emendamento, che non abbiate neanche provato a capire che cosa c'era dentro quella proposta e se era forse ragionevole dedicare un afflato afflato unitario a dei lavoratori che non sanno se torneranno a casa la sera dal lavoro. Anche perché - confesso che mi stupisce ho avuto la sensazione che la parola del Ministero del lavoro non fosse importante in questa discussione sulla legge di bilancio, altrimenti forse avrebbe dato delle motivazioni per non farlo. Ho sentito molto discutere in questo periodo di un tema giustissimo per il nostro Paese che si chiama natalità e che si chiama anche tenuta del sistema di *welfare* e del sistema previdenziale, in ragione del fatto che che il Paese per fortuna ha una maggiore aspettativa di vita, ma ha pochissime nascite. Eppure, ho visto solo provvedimenti che riguardano famiglie che hanno già dei figli. Forse, se dobbiamo occuparci di natalità, dobbiamo occuparci di costruire le condizioni perché altre famiglie provino a fare dei figli, perché altrimenti la situazione non si muove. *(Applausi)*. Vorrei ricordare a tutti noi che qualche giorno fa abbiamo analizzato - anzi ha analizzato l'Istituto - le ragioni delle dimissioni volontarie. Siamo di nuovo dinanzi al fatto che ci sono più di 40.000 lavoratrici che hanno dato le dimissioni perché non potevano conciliare la loro vita personale e il rapporto di lavoro. Anche qui c'è una piccola cosina che vi abbiamo proposto: perché non diciamo che per quelle lavoratrici, quando denunciano il fatto che non sono in grado di conciliare, possono avere una sede - sono le sedi degli Uffici regionali del lavoro - in cui provare a costruire con le aziende delle forme di flessibilità che permettano loro di continuare a lavorare? Altrimenti quella lavoratrice dovrà scegliere, un minuto dopo, se potrà fare un altro figlio oppure se non potrà più farlo. Ed è così che ammazziamo la prospettiva e la volontà delle lavoratrici e delle donne di essere madri. Lo stesso vale per i congedi paritari. Ci avete provato a dedicare un occhio? Avete provato a ragionare se dentro quella scelta c'era una risposta positiva che provava a redistribuire un carico del lavoro di cura che, se non si redistribuisce, rende sempre più difficile il nostro *welfare*? Abbiamo provato a ragionare e lo diciamo molte volte rispetto a questa manovra - sul fatto che guardare la prospettiva vuol dire anche guardare che cosa facciamo di un sistema produttivo industriale che è in grande difficoltà. Ilva di Taranto, Stellantis, oggi un *call center* di quasi 500 dipendenti in Calabria: ci sono migliaia di crisi aziendali, ci sono settori che sono stati strategici per il nostro Paese e che oggi non hanno una risposta. E non c'è una scelta dal punto di vista degli investimenti, ma non c'è una scelta neanche dal punto di vista della protezione di quei lavoratori di fronte ai processi di ristrutturazione e alle preoccupazioni che ci sono. Capisco che ci sia un giusto entusiasmo perché finalmente abbiamo dato una risposta ai lavoratori poligrafici. Vorrei dire che c'era un nostro emendamento che diceva quella cosa e, quindi, non capisco perché venga rinfacciata all'opposizione. Ma non ci sono solo i lavoratori poligrafici in questo Paese. Quando si danno risposte solo per alcuni settori e per altri non si danno, in realtà si determinano delle diseguaglianze e non delle risposte positive. *(Applausi)*. Ed è la cosa che vi dico sui lavoratori fragili. Capisco che volete far finta che il Covid non ci sia, che volete far finta che siamo tutti in salute e che non ci siano più problemi, ma - ahimè - ci dicono altre cose gli ospedali e le terapie intensive. E allora davvero mi domando: qual è la crudeltà che vi porta a pensare che quei lavoratori dobbiamo esporli al fatto che possano ammalarsi, ma anche qual è il risparmio che pensate di avere da tutto questo? Certo, non spenderete per fargli avere le condizioni di lavoro agile e le condizioni per poter rimanere a casa e non contagiarsi, ma spenderete quelle risorse in sanità, rendendo ancora più difficile un sistema sanitario cui continuate a tagliare le risorse. Ci sono delle cose che davvero non mi riesco a spiegare. Non me le riesco a spiegare, perché non sono delle domande che richiedono chissà quale ammontare di risorse; richiedono in realtà molto meno di quello che richiede il sogno del Ponte sullo Stretto di Messina, che non è necessario e che invece distoglie tante risorse che farebbero tanto bene a tante persone. Avete detto che ci sono grandi risposte per il lavoro. Vorrei dirvi che, per un lavoratore italiano, la busta paga di dicembre e la busta paga di gennaio saranno uguali. Un lavoratore italiano nel 2024 non avrà un euro in più di quello che ha avuto nel 2023 per vivere. Non gli avete aumentato la retribuzione: avete solo scelto che il cuneo continuasse a essere una norma che viene prorogata di tempo in tempo, per rivenderla ogni volta, rivenderla ogni volta, ma non aumentate le retribuzioni dei lavoratori. Lo dico anche rispetto al modo in cui state utilizzando i contratti nella pubblica amministrazione, dove non contrastate la precarietà - per carità - perché è bene che le amministrazioni locali non siano nelle condizioni di lavorare bene per il PNRR. Ma, nello stesso tempo, quei contratti contratti sono dovuti; non è una vostra libera iniziativa di soddisfare le condizioni dei lavoratori. *(Applausi)*. I contratti sono dovuti e voi dovreste saperlo, visto che avete esattamente usato i contratti di lavoro come arma per dire "no" al salario minimo. E allora aumentateli quei contratti di lavoro e, quando dite che ci sono organizzazioni sindacali che firmano contratti troppo bassi, vorrei dirvi: date uno sguardo alle pubbliche amministrazioni, date uno sguardo a quali appalti hanno e a quanto pagano per quelle retribuzioni. Vado a concludere, Presidente. Non parlo delle pensioni, su cui ci sarebbero molte cose da dire. Una cosa però credo sia necessaria: ci avete raccontato che voi sì che avreste mandato i lavoratori e le lavoratrici in pensione con quarantuno anni di contributi. I medici vi ringraziano, perché sono a quarantasei con il vostro provvedimento. *(Applausi)*. Ma vorrei chiudere su una cosa, perché oggi è una giornata strana. È una giornata in cui non si risponde ai lavoratori dell'Ilva di Taranto, ma in un tribunale di Roma arriva la sentenza dopo l'assalto alla sede della CGIL dell'ottobre 2021. Noi siamo contenti che ci sia stata giustizia, esattamente perché un giudice c'è. Ma vorremmo dire al Governo tramite lei, signora Presidente, e a tutto il Senato che troviamo un po' sconvolgente che in un anno in cui abbiamo trovato nuovi reati e pene aumentate, in cui sembrava che ci sarebbe stata qualunque forma d'ordine necessario, si possa fare il saluto romano in un'aula di tribunale per contestare una sentenza. Io mi auguro che si apra un'indagine su quello che è successo.

delusi per quanto è stato fatto nel disegno di legge sul *made in Italy* e adesso che si è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio. Parlare di turismo e di promozione significa parlare di infrastrutture, di sicurezza,

la manutenzione della galleria Passo del Lupo tra la Puglia e il Molise, che va avanti da quest'estate e non si sa se riaprirà quest'anno. I pendolari sono davvero allo stremo perché sono costretti a prendere l'autostrada, quindi aumentando i costi, o una strada provinciale interna in zone di montagna, che questo inverno sarà anche doppiamente pericolosa vista la possibilità di neve e ghiaccio. Vorrei quindi sollecitare il Governo e tutti i miei colleghi ad attenzionare una velocizzazione dei lavori di manutenzione, perché è impossibile continuare con continue interruzioni. Le autostrade sono impercorribili, i tempi sono davvero troppo lunghi e allora stanziamo fondi per la manutenzione delle strade, perché questo significa davvero parlare di promozione territoriale, di *made in Italy*, di turismo e quindi di benessere per tutti i cittadini italiani.

La seduta è tolta